La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 9 marzo. Nella seduta di oggi sarà discusso, fino alla sua conclusione, il decreto-legge sul contrasto all'emergenza Covid nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito, stabilendo che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama. L'ordine del giorno di oggi è inoltre integrato con il disegno di legge sull'agricoltura con metodo biologico, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale non sono stati presentati emendamenti. La prossima settimana sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge sostegni. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 9 marzo per l'esame del disegno di legge delega in materia di contratti pubblici e della relazione sulla domanda di autorizzazione sull'utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Siri. in sede di esame del provvedimento recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; alla Presidente delle Commissioni riunite 1a e 12a, senatrice Parente, di riferire sui lavori delle Commissioni. del disegno di legge n. 2542 la seduta pomeridiana di ieri e quella antimeridiana di stamattina. Sono state svolte le fasi dell'illustrazione, della discussione generale, delle repliche

date anche le numerose richieste di intervento per l'illustrazione e le dichiarazioni di voto. Conseguentemente, non è stato possibile terminare l'*iter* in Commissione con il conferimento del mandato ai relatori. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla senatrice Parente, il disegno di legge n. 2542, non essendosene concluso l'esame nelle Commissioni

quale l'Europa era centrale, quanto a importanza politica, in uno scenario delicato qual è quello del conflitto in Ucraina.

spinta a darsi una maggiore consistenza, sotto il profilo politico. Voi conoscete benissimo le mie posizioni rispetto all'Europa e all'Unione europea. Avendo messo in piedi un partito che si chiama Italexit, non ho una grande considerazione del progetto europeo o unionista, ma mi rifaccio e mi rimetto sulla scia delle vostre parole, anche per costruire un pezzo della questione pregiudiziale. Se infatti è vero che, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con l'abuso della decretazione d'urgenza; e se, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con le tante questioni di fiducia e i tanti voti di fiducia, è altresì importante richiamare lo scollamento che c'è tra la normativa italiana e quella europea e, quindi, con quell'Europa di cui continuate in un certo senso a invocare il rispetto e la costruzione. e la costruzione. Attraverso la decretazione d'urgenza è stata costruita praticamente tutta l'impalcatura normativa dell'emergenza Covid, ma a un certo punto anche qualche altro soggetto, l'Unione europea, stava tentando di dare una risposta normativa che rendesse omogenei che rendesse omogenei gli interventi dei Paesi membri dell'Unione europea. Tra questi vi è il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 953 del 2021. 2021. Proprio andando nelle pieghe di tale Regolamento, e in particolare dell'articolo 3, che, ai commi 1 e 7, vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino, tampone rapido o molecolare), ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico il certificato verde derivante dal tampone antigenico a quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione, dobbiamo capire che una cosa esclude l'altra: il *super green pass* o *green pass* rafforzato toglie uno dei tre elementi con cui finora abbiamo costruito un pezzo anche della nostra emergenziale vita quotidiana.

infatti, difficile riuscire a immaginare i giorni futuri e il periodo futuro stando ancora nella dinamica di una continua esibizione, di una continua ostensione, di un QR *code*, di un codice, di un *green pass*. È quasi come se avessimo sostituito i nostri nomi e le nostre carte d'identità con un quadrato magico. Penso che questo non sia in linea con l'addensante della Costituzione, che è ben più che la somma degli articoli, è un qualcosa che mette l'individuo al centro. Proprio alla luce del citato Regolamento, ritengo che il decreto che andiamo a discutere sia scollato, sia in antitesi, sia penalizzante. Da qui, invito i colleghi a fare una riflessione su che cosa vogliamo scegliere, a questo punto. Vogliamo battere o meno la via della soluzione italiana, nazionale, per uscire dall'emergenza, come mi sembra nello spirito di quest'Assemblea?

arriva dentro il Regolamento che, tra le norme e gli atti normativi dell'Unione europea, è il più forte e il più vincolante in tutte le sue parti. Allora, perché continuiamo ad andare avanti su una strada che non non impatta più sulla vita di oggi, perché non siamo assolutamente più nell'emergenza di un tempo, da un punto di vista normativo, va a sbattere con quanto indica il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea? È un *green pass* rafforzato che rischia di essere indebolito proprio alla luce di questa conflittualità. Mi rimetto anche a un altro ordine di considerazioni, forse un po' più politico, ma che sta ancora una volta dentro la Costituzione, che non prevede in alcun modo la discriminazione tra gli individui.

che è anche bello che le piazze italiane si stiano riempiendo al grido di: no guerra, sì pace. Ben vengano tutta questa confluenza e tutta questa partecipazione larghissima di persone. Sono sicuro che in quelle piazze si troveranno persone che magari non avrebbero partecipato insieme a manifestazioni contro il *green pass*. E potrebbe accadere che il sabato e la domenica vadano insieme in piazza a dire no alla guerra, e poi, il lunedì, qualcuno sarà discriminato, perché non in possesso del *green pass* rafforzato, e quindi sarà escluso dal lavoro, da un suo diritto costituzionale. Ovviamente, mi auguro che lo scenario di guerra vada a concludersi nel più breve tempo possibile. Ma, se così non fosse, com'è sacrosanto il diritto dei cittadini di dire no alla guerra, lo è altresì il fatto di denunciare la paradossale situazione per cui mi ritrovo a dire no alla guerra e sì alla pace, a stare insieme in piazza con tante altre persone, e magari il lunedì a non poter andare a lavorare, perché sono stato penalizzato.

nel mondo della scuola, delle Forze dell'ordine, della sanità, e quindi nelle tre categorie professionali che sono state segnalate e marchiate dall'obbligo vaccinale, non può avere diritto a tornare sul posto di lavoro? quantomeno a dire sì o no su una pregiudiziale che vi consentirebbe di esprimervi. So che dentro quest'Aula ci sono sensibilità politiche politiche diverse e qualcuno avrebbe voglia di smarcarsi e di dire basta a quest'emergenza trascinata a fatica. Allora, siccome non siamo un QR *code* e siamo tutti ben consapevoli delle discriminazioni che possono nascere e si possono alimentare, vi invito a prendere in considerazione proprio questo aspetto. Vogliamo e volete essere pienamente europeisti oppure volete in qualche modo difendere soltanto l'attività del Governo? È questo il succo della questione pregiudiziale che rimette il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo proprio al centro: quello è il pallone con cui dobbiamo giocare.

Venire oggi a dire al Parlamento che non deve convertire un decreto-legge, che peraltro scade fra sei giorni, è un inutile tentativo di ostruzionismo, di *filibustering*.

vedrà che i decreti-legge in tema di contenimento del Covid e della crisi economica a esso legata sono stati per l'esattezza 42, dall'inizio della crisi ad oggi. Tutti i provvedimenti sono stati presi nell'alveo del diritto europeo e della Costituzione italiana, garantiti dalla firma autorevole del garante della Costituzione, il presidente Mattarella. C'è stata un'ansia normativa che ci auguriamo di non vedere mai più, ma che assolutamente giustifichiamo, in quanto dovuta all'evolversi di eventi imprevedibili e incontrollabili.

La scienza all'inizio della pandemia non sapeva chi fosse il nemico né come affrontarlo, per cui la prudenza sua e dei comitati scientifici che consigliano il Ministro della salute ha richiesto la necessità di adattare via via i provvedimenti *in* *itinere*. La stessa prudenza è stata presa nell'adottare atti normativi in favore degli italiani. Se però non ci fossero stati tutti i provvedimenti emanati, oggi non saremmo a quasi il 90 per cento di vaccinati e non avremmo salvato migliaia e migliaia di vite umane. Ricordo che il primo anno della pandemia, quello che ci ha visto quasi senza difese, ha fatto 130.000 morti. Il numero dei deceduti è poi calato grazie alle misure prese nello stato di emergenza. La gestione tecnico-scientifica della pandemia e quella dei provvedimenti ad essa collegata poteva essere fatta con maggiore razionalità? Forse sì, ma la prudenza ha rallentato le diverse varianti del *virus* e ha salvato migliaia di vite, soprattutto dei soggetti più deboli, portandoci ora ad avere maggiore consapevolezza di chi è il nemico, di come muta e di come possiamo affrontarlo. Quello che conta oggi è che, nel momento in cui stiamo affrontando l'argomento e approvando il provvedimento al nostro esame, siamo entrati in uno stato nuovo dell'emergenza Covid-19. Siamo fuori dall'emergenza: sì, siamo nella fase finale e, se anche ricominciasse una nuova variante, abbiamo oramai informazioni sufficienti per affrontarla senza chiudere nuovamente tutto e direi anche senza imporre nuove restrizioni sanitarie che non siano di buon senso. La durata del *green pass* è cambiata diverse volte, è così; quella del *super green pass* ora è finalmente illimitata. Oggi abbiamo alcune certezze: i vaccinati - quasi il 90 per cento della popolazione adulta hanno contribuito certamente a rallentare, ma non a fermare la circolazione del virus. Sicuramente sapremo affrontare nuove epidemie o pandemie con gli strumenti più adeguati: oltre ai vaccini e agli eventuali richiami, ne abbiamo di nuovi, sempre più specifici; abbiamo altre cure e protocolli di cura da seguire, che si sono dimostrati efficaci. Ribadiamo la nostra fiducia nelle vaccinazioni, ma oggi siamo confortati dal fatto di avere anche altri percorsi sanitari da far seguire a chi non possa o non voglia vaccinarsi. quindi più distinguere tra buoni e cattivi, perché così facendo abbiamo dato voce ai cattivi maestri, tra i quali i no vax e i no mask,

che hanno subito pesanti perdite. Lo dobbiamo anche agli altri settori produttivi che hanno subito un contraccolpo straordinario. Lo dobbiamo ai lavoratori, che devono poter tornare a lavorare in tranquillità. Ci auguriamo che i nostri ragazzi possano tornare a frequentare la scuola sempre in presenza. I genitori di ragazzi disabili - così come prevede il decreto-legge - nel settore privato potranno usufruire dello *smart working.* Ritengo quindi, che gradualità e buon senso debbano essere le nuove parole d'ordine che segnano la fine del periodo di emergenza durato due anni. Con prudenza, cautela e responsabilità, ma senza allarmismi, dobbiamo e possiamo contrastare il virus e le sue varianti, tornando però in modo graduale e convinto alla normalità, peraltro segnata da tensioni e conflitti, che ci devono indurre a lavorare tutti per proporci come messaggeri di pace. In considerazione di quanto detto, il Gruppo Forza Italia invita a un voto contrario alla questione pregiudiziale È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

in merito ai provvedimenti che sono stati fin qui adottati. Mi riferisco soprattutto all'efficacia della campagna di vaccinazione e alle modalità con le quali è stata condotta.

sia ai comportamenti diligenti della gran parte degli italiani sia all'efficacia della campagna di vaccinazione. Lo dobbiamo cioè ai vaccini, che hanno aumentato le nostre resistenze

Personalmente, Presidente, signori colleghi e colleghe, non sono un fautore degli obblighi. Negli oltre quarant'anni di esperienza professionale e di vita da medico, seppur condotta da medico ospedaliero, ho dedicato davvero molto tempo alla prevenzione, andando incontro alle carenze dell'assistenza territoriale che sono ben note e che cercheremo di sanare di sanare con l'attuazione dei provvedimenti del PNRR. Ci siamo dedicati tanto negli ospedali alla prevenzione e, come me, tanti colleghi si sono resi conto di quanto sia importante l'adesione spontanea individui, che si può ottenere a seguito del dialogo e di una corretta informazione. Bisogna convincere le persone dell'efficacia delle pratiche mediche, cosa che purtroppo non sempre è avvenuta, a causa di una comunicazione che spesso ha prestato più attenzione all'*audience* che alla vera e propria opera di informazione.

Ciò che mi dà da pensare è che difficilmente si sarebbero raggiunti i traguardi odierni, noti a tutti, se non fossero state introdotte determinate misure.

constatare come le persone credano all'efficacia e alla validità delle cure mediche e delle terapie chirurgiche e si affidino a noi medici, sapendo che risolveremo la grande maggioranza dei loro casi, perché ovviamente pratichiamo una medicina basata sull'evidenza, che viene dalle esperienze professionali di tutti e ci mette in condizione di raggiungere i migliori risultati.

Mi ricollego al discorso di prima: forse bisogna rivedere le modalità di informazione e di scambio e bisogna parlare con le persone, proprio per evitare che si formino compagini tipo pro vax, no vax o pro scienza, contro la scienza. Questo sicuramente non fa bene alla società.

tutta la specie umana e rivedere alcune nostre abitudini. A questo proposito vorrei fare una precisazione e mi rivolgo anche ai decisori politici:

della ventilazione negli ambienti chiusi per ridurre fortemente le possibilità di contagio. Mi auguro quindi che il decisore politico introduca dei provvedimenti che possano facilitare e aumentare la ventilazione negli edifici pubblici e privati. concludo affermando che tutte le misure sono passibili di una revisione al fine di migliorarne l'efficacia. La scienza medica lo fa periodicamente, più volte nel corso dell'anno: vi sono società internazionali preposte a questo, che rivedono le linee guida che ispirano i nostri comportamenti e i protocolli medici. Bisogna sempre adattare i provvedimenti alle nuove circostanze e non vi è motivo di ritenere che, anche nel prossimo futuro, non possano essere modificati i provvedimenti sin qui adottati,

Aspettare ancora non ha senso: sono provvedimenti e misure che erano inutili e dannosi, per cui prima li togliamo e meglio è. Stiamo facendo un danno al Paese: ci sono cittadini che non hanno non hanno più diritto al lavoro e non hanno mezzi di sostentamento, e noi dobbiamo immediatamente far venir meno tutto questo. Vi invito quindi a riflettere: se voterete a favore di questa questione pregiudiziale, tutti i divieti, gli obblighi e la burocrazia ormai inutile verranno meno. Se invece voterete contro, vi renderete complici di ulteriori sofferenze e dovrete risponderne alle migliaia di persone che in questo momento sono a casa senza lavoro, o costrette a ottemperare a obblighi vaccinali che non vogliono e che comunque in questo momento non sono più attuali.

Ci apprestiamo a convertire in legge un decreto-legge del Governo, le cui disposizioni appaiono già fuori contesto e per molti versi non perfettamente allineate con le più attuali evidenze scientifico-sanitarie. Le morti da Covid costituiscono una straziante e lacerante realtà e, al di là di qualche ragionevole dubbio sulla correttezza e accuratezza della relativa stima, restano comunque tante e troppe; ugualmente, le morti e gli eventi avversi da vaccino sono verosimilmente sottostimati, per difficoltà di vario tipo nel denunciare e comprovare l'eventuale correlazione tra causa ed effetto. Non credo che possa esserci una morte più degna di considerazione di un'altra; non credo che ci possano essere paure più nobili di altre. Non ci sono verità assolute e altre da denigrare o deridere a prescindere; ci sono pensieri, riflessioni e parole di persone più o meno sensibili, preparate e attente e più o meno capaci di argomentare un pensiero oggettivamente critico. La scienza e i vaccini hanno da sempre reso un servizio prezioso alla collettività e alla salute pubblica, ma le contraddizioni di alcune misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del SARS-CoV-2, che ha a sua volta favorito l'innescarsi di un effetto indotto, non hanno facilitato un dialogo e un confronto realmente persuasivo. Di contro, hanno alimentato antagonismi, contrapposizioni e dispute ideologiche, nel cui solco attecchiscono e si rafforzano la cultura del sospetto, la malafede e l'ignoranza. La pandemia ha prodotto vicende tristi e dolorose in termini non solo sanitari, ma anche economici, ha preso tutti alla sprovvista. Oggi, però, una maggiore consapevolezza degli eventi ci impone di non essere spettatori inermi e acriticamente passivi rispetto a una realtà che va tenuta distinta dalla spettacolarizzazione mediatica. Traendo insegnamento dall'esperienza vissuta e rendendo merito al sacrificio di tutti coloro che si sono fatti parte attiva in questo difficile percorso comune, la politica ha il dovere di porsi con piglio costantemente critico e responsabile, accogliendo ogni voce, anche quella apparentemente più insensata, con la forza di chi, in maniera equilibrata e mai faziosa, è chiamato a operare nelle scelte con atteggiamento fiducioso, ma non fideistico, perché la stessa scienza ci ha dato prova che nulla può mai essere osservato in modo assoluto. Domando a quest'Assemblea se non sia giunto il tempo di cambiare approccio strategico rispetto a un quadro epidemiologico in favorevole divenire, in favorevole divenire, concentrando ogni sforzo su quella parte di sanità, prima fra tutte la medicina territoriale (vero argine di ogni epidemia da virus), che richiede interventi strutturali e non più emergenziali, rafforzando i protocolli di sicurezza nei luoghi sovraffollati e negli ambienti di lavoro e, non da ultimo, incentivando il lavoro agile. Il certificato verde - o *green pass* che dir si voglia - la cui asseverata funzione, in concreto e senza ipocrisia di sorta, è stata ed è fondamentalmente quella di indurre alla vaccinazione le frange più riottose, con qualche qualche imbarazzo sul fronte dei presidi costituzionali, tende a essere ormai percepito come un ingiustificato e pervicace tentativo di continuare ad utilizzare le maniere forti. Tuttavia, in un contesto globale in cui la reale e contingente emergenza è rappresentata da un aumento incontrollato del costo della vita e da un tessuto economico e produttivo ancora troppo fragile, l'eccesso di prudenza può essere scambiato per accanimento ingiustificato, ingenerando ulteriori e pericolose tensioni. Mi pare di capire che sia giunto, infine, il momento di superare, con spedita e non equivoca gradualità, la fase delle restrizioni, guardando con fiducia alle scelte operate anche da altri Paesi e non dimenticando e non dimenticando che il lavoro, l'istruzione e la socialità in genere sono diritti che vanno tutelati e garantiti al pari della salute. Dobbiamo evitare di prestare il fianco, con le nostre scelte politiche, ad atteggiamenti anche indirettamente o inconsciamente discriminatori, aggravati o addirittura causati da un approccio non sempre serenamente obiettivo, perché contaminato dall'esigenza di trasformare in spettacolo persino il dibattito scientifico. Non possiamo permetterci di penalizzare la ripresa economica, adottando misure che sono state necessarie, ma che devono rappresentare un estremo rimedio. Il Paese e l'intrapresa economica vanno sostenuti, ma soprattutto hanno bisogno di correre sulle proprie gambe, senza vincoli che non siano davvero giustificati. È opportuno dunque analizzare i dati reali, gestiti in maniera corretta, trasparente e indipendente, senza pressioni o ingerenze sulla scienza e sulla politica per avvantaggiare l'una o l'altra fazione o, peggio, per trarre un indebito profitto. I cittadini vanno stimolati al dialogo e al confronto, non assoggettati all'imposizione e la politica deve saperlo fare, assumendosi le proprie responsabilità, giammai delegando ad altri le decisioni che le competono. Nel rispetto dei canoni di adeguatezza e ragionevolezza, è necessario pertanto riportare con coraggio, determinazione, forza e fiducia il tessuto economico, sociale e produttivo verso la normalità. Solo così si potrà rendere un buon servizio alla collettività, pacificando gli animi e superando ogni insicurezza e timore.

decoro al dibattito che segue questi provvedimenti, che arrivano dal Governo in modo difficile da aggettivare. Per l'ennesima volta, arriviamo a esaminare in Aula un provvedimento importantissimo, che incide sulla vita quotidiana degli italiani in modo stringente e tale e tale da condizionarne non solo gli atteggiamenti, ma anche il vivere quotidiano e persino il mangiare. E chiariremo poi perché dico questo. Ci arriviamo ancora una volta senza relatore vedremo che cosa accadrà rispetto alla possibilità di discutere in Aula gli emendamenti. Questa mattina in Commissione, ovviamente, per il sovrapporsi degli orari e dei calendari non è stato possibile affrontare gli emendamenti, non abbiamo neanche esaurito l'esame

Gruppo Fratelli d'Italia che, come stamattina e come in altre occasioni - vorrei dire come sempre, da quando il Governo si è insediato garantisce al Parlamento almeno un minimo di decoro. Lo stiamo facendo anche in queste condizioni, sapendo che parliamo a beneficio del Resoconto Lo facciamo a prescindere da ogni altra considerazione, perché evidentemente abbiamo ben chiaro quali sono il nostro ruolo e la nostra responsabilità e rispondiamo, come sempre, agli italiani. In questo provvedimento ci sono - come ho detto - numerosi passaggi e mille incongruenze.

e lo facciamo, evidentemente, a beneficio di quello che è accaduto. In una condizione normale, un Governo normale avrebbe invece dovuto cambiare questi provvedimenti e renderli compatibili con la conversione dell'Assemblea, cosa che si è sempre fatta e che evidentemente non trova più spazio negli atteggiamenti e nelle posture - per usare un termine che ho sentito ieri - di questo Governo che si atteggia a

il più importante - a mio avviso - è il riconoscimento della parte alimentare dello stipendio.

riconoscere la componente alimentare insopprimibile dello stipendio di chi è sospeso dal lavoro perché non ha provveduto alla vaccinazione, fare un esempio - questa parte alimentare dello stipendio viene riconosciuta ai mafiosi, agli assassini o a tutti coloro i quali - dipendenti pubblici sono sospesi dal servizio in attesa del percorso processuale che li vede imputati per reati gravissimi, anche odiosi. a quelli vengono riconosciute l'indennità e la parte alimentare dello stipendio, ma a coloro i quali sono sospesi dal lavoro e dallo stipendio perché non hanno provveduto alla vaccinazione non viene riconosciuta la parte alimentare dello stipendio. È così, Presidente, non viene riconosciuta. *(Applausi)*. C'è gente che non arriva a poter garantire alla propria famiglia la spesa alimentare. Mi sembra di vedere Mi sembra di vedere l'incredulità negli occhi dei colleghi che ascoltano - pochi a dire il vero - ma vi garantisco che questo accade: esistono anche emendamenti della parte politica della Presidente che hanno tentato di far capire al Governo che non si può continuare così.

avete fatto questa considerazione banale? Vi rendete conto che quello è un vaccino che ha la stessa tecnologia e le stesse risultanze di effetto e di validità

Quindi, che cosa faremo con questa gente? Li rivacciniamo di nuovo oppure li lasciamo senza *green pass*, con tutto quello che comporta? Che cosa accadrà a questa gente che arriva da quel territorio di guerra e sopraffazione?

il vaccino di tutti i coloro i quali non si erano vaccinati finora perché non si fidavano o non si affidavano a quello che gli avevamo raccontato riguardo alla validità dei vaccini fino a questo momento utilizzati. il vaccino Novavax è un fallimento, nel senso che tutte le Regioni l'hanno messo a disposizione, ma non c'è accesso a questo vaccino; e ormai è registrato ampiamente. Accade quindi, colleghi, che quello che si doveva fare fin dall'inizio, ancora oggi non lo stiamo facendo; ancora oggi pensiamo di voler costringere la gente a vaccinarsi anziché convincerla. E come è possibile convincere la gente a vaccinarsi, collega Sileri? È possibile attraverso i medici di medicina generale. Recentemente, abbiamo tenuto un'audizione in Commissione con i rappresentanti sindacali dei medici di famiglia, i quali hanno dichiarato che nessuna Regione ha messo a disposizione dei medici i tabulati dei loro assistiti che non sono coperti dal vaccino; non c'è stato *feedback*, non c'è stata collaborazione, non c'è stato coinvolgimento della figura principale a cui il cittadino deve affidarsi. affidarsi. A chi si deve affidare il cittadino? Alla Gruber e a «Otto e mezzo»? A chi si deve affidare il cittadino se non al suo medico di famiglia? Ebbene, i medici di famiglia sono stati sempre, costantemente,

finestre. Se questo è accettabile in un Paese civile e moderno, lo lascio considerare a voi. Abbiamo approvato degli emendamenti che riguardano la possibilità di adeguare le aule

L'ha detto il Presidente della Repubblica. Non lo dice il povero senatore di campagna, ma l'ha detto il Presidente della Repubblica. Bisogna dare un taglio e, se non lo fa la Presidenza del Senato, mi domando e vi domando: chi lo deve fare? Chi è che deve richiamare ognuno al senso di responsabilità consono al proprio ruolo e a esercitare fino in fondo le proprie prerogative, come prevede il percorso costituzionale, e non oltre? Stiamo

vecchi, che risalgono al 5 novembre e al 12 dicembre 2021. Il decreto, per sua natura, ha una durata provvisoria quindi, non c'è assolutamente necessità di convertirlo in legge, laddove le evidenze di questo periodo ci dicono che è assolutamente insensato farlo. È insensato, perché è un accanimento contro persone che hanno deciso di non vaccinarsi, scientemente, o perché non lo possono fare per ragioni di salute o perché non si sentono tutelate da questi prodotti, che non hanno seguito un *iter* sperimentale regolare. E ne hanno tutto il diritto, perché glielo riconoscono le convenzioni internazionali: glielo riconosce la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea, glielo riconosce la Convenzione di Oviedo; glielo riconosce anche il Regolamento 2021/953, che è un atto sovraordinato rispetto anche al nostro ordinamento, perché è un regolamento europeo e, quindi, direttamente

Questi prodotti vengono imposti anche a persone che hanno una immunizzazione più aggiornata rispetto a quella che può offrire questo vaccino. Non si può, infatti,

i casi di effetti avversi in Europa e sono quasi 40.000 i decessi correlati o avvenuti in prossimità della somministrazione di detti prodotti. Con queste premesse si vuole confermare, convalidare e trasformare in legge un decreto che praticamente conferma un obbligo vaccinale per le persone over cinquanta, fuori da ogni parere del Comitato tecnico-scientifico, che non si è nemmeno espresso, perché non può esprimersi, perché questo decreto non ha alcun fondamento sanitario. In premessa esso dice il falso, perché nessuna emergenza sanitaria può essere assolutamente contenuta con i provvedimenti previsti in questo decreto. L'emergenza sanitaria è finita ovunque, ma rimane in Italia fino al 31 marzo. Questa è un'assurdità solo nostra, fatta perché bisogna accanirsi per affermare un

ci dicono che questi prodotti alla fine non sono efficaci a contenere né i contagi, né le ospedalizzazioni e nemmeno i decessi per Covid. Ciononostante, si procede sulla stessa linea fino al 15 giugno, secondo voi e secondo anche tutti quelli che hanno parlato. È assurdo: ci sono dei senatori della maggioranza che si sono espressi contro, hanno già detto che il decreto-legge è fuori luogo e fuori tempo. Eppure, oggi che faranno? Voteranno la fiducia? Come ieri hanno votato per la risoluzione di maggioranza, pur dichiarandosi contro la guerra? Confermeranno così una linea folle che ci sta portando simultaneamente a una guerra,

economica gravissima che riguarda l'economia dei territori, l'economia reale. Nonostante ciò, si continua a voler tenere in piedi un Governo che sta facendo solo danni all'Italia e a

noi siamo un intero Paese in balia di una maggioranza che, come un automa, non fa altro che approvare provvedimenti

di un'intera Nazione? Quale senso di responsabilità state esibendo? Voi come maggioranza volete tenere in piedi questo Governo e questa legislatura. Ma a cosa serve tenere in piedi una legislatura che sta legiferando in questo modo? Il ruolo del Parlamento è stato completamente cancellato. Ci sono addirittura colleghi che oggi non potranno votare, così come non hanno votato l'altra volta, a causa del

che non ha alcun valore costituzionale e limita il loro mandato attraverso un atto burocratico amministrativo che in questi luoghi è inammissibile. Quando siamo stati eletti, parlamentari hanno dovuto imparare a memoria i nostri volti, perché noi non dovevamo esibire neanche un documento di riconoscimento, e adesso imponete a tutti i parlamentari l'esibizione di una tessera che non attesta nulla, non attesta alcuna sicurezza sanitaria: attesta solo l'obbedienza cieca e folle a norme che non hanno alcun senso, che sono soltanto il simbolo di un potere autoritario che state imponendo. Avete trasformato la nostra Repubblica parlamentare democratica fondata sul lavoro in una Repubblica autoritaria fondata sull'emergenza.

Qualche punto di contatto critico ce l'abbiamo tutti per l'affollamento con cui i provvedimenti si stanno sovrapponendo gli uni agli altri per cui, quando arrivano alla nostra attenzione, in certi casi alcune delle norme che contengono sono già superate; la qual cosa dà una sensazione di estraneità. Non voglio entrare nel merito della lettura puntuale del decreto-legge per ricavarne gli elementi che avrebbero potuto essere per così dire migliori. Voglio concentrarmi su due obiettivi importanti, il primo come abbiamo ripetuto tante volte in questa legislatura - è il diritto alla salute. Mai come in questa legislatura abbiamo saputo, voluto e potuto porre il diritto alla salute al centro del dibattito generale. Lo abbiamo voluto fare in una dimensione molto particolare, che è il diritto alla prevenzione.

si era fatta un'operazione di prevenzione attraverso la vaccinazione di questa portata. Questo credo che vada a onore di coloro che l'hanno programmata,

la tutela della propria salute e la tutela della salute delle persone che ci stanno accanto. Questa è la grande forza della prevenzione: sapere che non sto perseguendo

Proprio per questo, colleghi, Presidente, membri del Governo, per l'importanza e per l'enfasi che è stata messa in questa legislatura sul diritto alla salute ottenuto attraverso la prevenzione - un approccio molto alto come sguardo sulla salute pubblica - mi auguro che, per quella ricchezza che ci conferisce il sapere traslazionale, questo stesso atteggiamento possa essere proiettato su tante altre patologie. altre patologie. La concentrazione dell'interesse di tutto il sistema nei confronti della lotta al Coronavirus, infatti, ha fatto sì che abbiamo lasciato nell'ombra,

a volte lo fa con un'attenzione così minuta, così puntuale, così precisa, così difficile anche da governare, proprio per la quantità e la qualità delle eccezioni che prende in considerazione, che - dobbiamo riconoscere - è la risposta a una critica che - in modo direi condiviso - abbiamo mosso tutti rispetto al rischio che noi ritenessimo di poter soddisfare il diritto dei bambini all'istruzione soltanto attraverso la famosa didattica a distanza. Per evitare la didattica a distanza si è moltiplicata l'attenzione alla prevenzione all'interno della vita scolastica,

la qualità della vita e la salute delle persone che andavano a lavorare. E, ancora una volta, l'abbiamo fatto cercando di spezzare il circuito in cui la cultura del nostro tempo ci sospinge continuamente, che è il diritto individuale, ponendo in evidenza il dovere sociale. Quindi, nei posti di lavoro abbiamo alzato il livello della sensibilità rispetto all'obbligo di una vaccinazione che fosse a tutela delle persone fragili.

della salute di chi ci sta accanto, senza per questo rinunciare a quella straordinaria esperienza umana che è per tutti noi la possibilità

Il lavoro significa molto, come grande laboratorio di esperienza umana. Chi è stato a casa nei famosi mesi del *lockdown* duro sa quanto era difficile realizzare un lavoro che conservasse tutta la sua dimensione di ricchezza umana, di collante della coesione sociale. Il decreto-legge in esame, nella misura in cui sottolinea il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro, stabilisce una sorta di triangolazione molto importante, nella quale si inquadra tutto il nostro sistema di vita, personale e sociale, privato e pubblico; tutta la nostra vita è sfaccettata su questi tre grandi diritti.

di trasferimento di competenze, di sensibilità, di possibilità di imparare a dialogare con gli altri. Siamo sottraendo il bambino a quella forma di isolamento

La conoscenza mediata dal video, come il lavoro mediato dal video, possono in certi momenti essere una risposta positiva; possono contribuire a risolvere alcuni problemi, ma non possono sostituire le esperienze di realtà di cui ognuno di noi ha bisogno.

non intervengo quasi mai in Aula, perché ascolto e mi faccio un'idea di tutte le cose di cui discutiamo e spesso sono d'accordo o in disaccordo con quello che viene detto. Oggi però devo farlo, perché la medicina mi ha salvato la vita più volte. Per fortuna sono vaccinato e per fortuna c'è stato un intervento celere della medicina per creare i vaccini

mano. Ovviamente empatizzo e conosco benissimo tutte le difficoltà che hanno incontrato le persone, le famiglie, i ragazzi, i lavoratori; difficoltà sostanziali che hanno messo a dura prova tutti; comprendo quindi anche i toni. Come diceva la collega Binetti poco fa, abbiamo avuto interventi anche pesanti, difficili,

e di un lento ritorno alla normalità. Parlo di lento ritorno alla normalità, perché bisognerà comunque prestare attenzione a quello che faremo, a dove andremo e a come ci comporteremo. Dovremmo avere imparato tante cose da questo periodo sui dati scientifici e ospedalieri, sulla situazione reale dei contagi, soprattutto sulle strutture mediche che sono fondamentali per la salute di tutti, e non di qualcuno. si tratta di un intervento con delle cose positive. No, assolutamente, perché questa emergenza lunga due anni ha evidenziato tutte le carenze della nostra società. Questa situazione di emergenza ha evidenziato carenze nella sanità, nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e potrei andare avanti

al signor Sottosegretario: stiamo aspettando dal 2019 i decreti attuativi del Registro nazionale dei tumori, che è fondamentale per la vita di tutti.

Oggi invece la situazione qual è? La gente non ha potuto avere l'unica cosa che - per esempio - si può fare contro il cancro, che è controllarsi.

perché non ci sono stati i controlli, perché i reparti erano pieni, perché c'era il Covid. Quindi, pensiamo e riflettiamo bene su quello che diciamo e su quello che è successo sotto i nostri occhi. In questo periodo abbiamo visto le persone scagliarsi l'una contro l'altra - io sono no vax, io sono sì vax, per me è tutto finto, io ho paura, eccetera - senza rispettare più niente e nessuno, urlando e insultando chiunque. avvenuto mentre il mondo andava in rovina e avrebbe richiesto maggiore unione e umanità, come vediamo anche oggi. Torniamo ai vaccini.

a me personalmente e a migliaia di persone, anche in questa sede, in estrema e drammatica difficoltà, ci hanno aiutato e salvato la vita dei supereroi che oggi chiamiamo infermieri, OSS, dottori, operatori *(Applausi)*: insomma chiunque abbia messo a rischio la propria vita per salvare la nostra, quotidianamente, mettendo a rischio anche la propria famiglia. Questo hanno fatto quelle persone. C'è chi gioca su questo ed è una cosa vergognosa, secondo il mio punto di vista. Credetemi: non per cattiveria, ma chi non l'ha vissuta non può capire tutto questo. Un ultimo pensiero: ci siamo trovati ci siamo trovati di fronte all'obbligo di ridefinire noi stessi e chi siamo, nelle relazioni obbligatoriamente deprivate, assenze scoperte o riscoperte, presenze mai valutate prima o poco osservate nell'interezza, tante parti del sé che hanno avuto modo di emergere e, quindi, sono state messe a disposizione di un'elaborazione personale e intima. Ritroviamo il sé e ritroveremo un nuovo noi. Mi avvio alle conclusioni, Presidente, con un semplice invito. Apriamo le menti e i cuori; impariamo qualcosa da questa difficile lezione, appresa a forza negli ultimi anni, e rendiamo omaggio al grande sacrificio fatto da tutte le famiglie, dai parenti, dagli amici e da tutti i cari persi in questo periodo, facendo vedere loro che oggi forse - e dico forse - siamo sulla strada per essere migliori.

l'Italia ha sempre dato una buona prova nel contrasto alla pandemia e anche le scelte assunte da questo Governo sono state molto importanti: pensiamo semplicemente al modo in cui hanno permesso di gestire la terza ondata, rispetto ad altri Paesi. Adesso però siamo in una frase completamente diversa: la quarta ondata non ha fatto particolari danni, in parte grazie ai vaccini e in parte grazie alle misure introdotte con il decreto-legge al nostro esame, quando c'era il rischio di avere milioni di italiani in casa. Non a caso tutti i Paesi europei stanno dismettendo le misure emergenziali, con l'idea di tornare, nel giro di poche settimane, alla piena normalità. Per queste ragioni fa un certo effetto dover convertire oggi un decreto-legge che aveva senso i primi giorni di gennaio, ma che lo ha molto meno oggi, soprattutto se da parte del Governo non arriva un chiaro messaggio sull'allentamento delle principali misure. Il nostro Gruppo è stato tra i primi, nel maggio 2020, a chiedere un allentamento, differenziando le Regioni in base al numero dei casi. Siamo stati i primi, un anno fa, a dire che la sperimentazione del certificato verde in Alto Adige era un modello per riaprire in sicurezza i luoghi chiusi siamo stati i primi, lo scorso autunno, a chiedere misure più stringenti, seguendo il modello 2G austriaco, per spingere sulle vaccinazioni; così come in alcuni frangenti abbiamo chiesto espressamente al Governo di introdurre l'obbligo vaccinale. Questo per dire che non abbiamo mai avuto un approccio pregiudizievole e non ci siamo mai iscritti alla fazione degli aperturisti o dei favorevoli alle chiusure, ma abbiamo sempre ragionato in base alla situazione reale e lo stesso facciamo anche adesso. Non ci sono più particolari ragioni per tenere in vita tutta una serie di restrizioni, dopo la fine dello stato di emergenza. Non so se davvero siamo fuori dal Covid, ma quel che è certo è che, nei mesi più caldi, il virus rallenta la sua corsa: l'ha fatto già nel 2020, figuriamoci adesso che siamo quasi tutti vaccinati e che 10 milioni di italiani hanno già contratto il virus. Dobbiamo alleggerire l'uso del *green pass*, eliminandolo per alcuni luoghi e tornando a quello base per tutti gli altri. Possiamo sostituire le mascherine ffp2 con quelle chirurgiche nei luoghi al chiuso, se non abolirle completamente questa estate. Dobbiamo fare soprattutto questa riflessione per le scuole: in età pediatrica - come ha detto anche il Comitato tecnico-scientifico - le ffp2 sono inadatte alle capacità polmonari dei bambini. Dobbiamo togliere tutte le limitazioni agli eventi, anche perché - come vediamo sui campi di calcio - la capienza ridotta porta non al distanziamento tra le persone, ma a una loro concentrazione in alcuni settori dello stadio. Dobbiamo fare una seria riflessione sulla quarantena, nell'idea che, se davvero il virus sta assumendo caratteristiche endemiche, va trattato come tale. Possiamo fare tutto questo e nel frattempo insistere nella campagna vaccinale, nella speranza che il nuovo vaccino Novavax aiuti a convincere qualche altro scettico.

sembra aver appannato l'impatto della pandemia. Eppure, sono due anni e oltre che il mondo e il nostro Paese sono stati e sono attualmente impegnati nella lotta contro il virus.

il Governo è impegnato a facilitare un percorso sanitario per la popolazione ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro Paese di origine, in particolare per le famiglie che già generosamente ospiteranno familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, sia nelle zone di guerra. È purtroppo scientificamente provato che le guerre peggiorano le condizioni di salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente quelle infettive. È purtroppo la storia delle pandemie. Già molte Regioni si stanno attrezzando per vaccinare le persone che arriveranno in Italia. Ricordiamo che l'Ucraina, purtroppo, purtroppo, è uno dei Paesi a basso livello vaccinale: soltanto il 33 per cento della popolazione è vaccinata con due dosi. Dico questo non per fare terrorismo, ma per prevenire anche la diffusione del del Covid-19, che non è sparito, e soprattutto per proteggere e fare tutto quello che dobbiamo per non diffondere il Covid-19 intanto nella popolazione ucraina. Dalle immagini che ci arrivano vediamo che tante persone sono

siamo particolarmente soddisfatti che questo ordine del giorno sia stato approvato. Tornando alla situazione del

I colleghi ricordavano che oltre il 90 per cento della popolazione è vaccinata, per cui è innegabile che il popolo italiano, giustamente, abbia aderito alla campagna di vaccinazione. E anche le risultanze del *green pass* base e del *green pass* rafforzato sono sotto gli occhi di tutti nel calo della curva epidemiologica. Naturalmente,

di emergenza. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli e coscienti che in realtà non abbiamo ancora una deflessione completamente verticale dell'impatto della pandemia. pandemia. Anche il nuovo vaccino magari ci aiuterà a convincere coloro che non si sono ancora avvicinati alla vaccinazione e si fa presente che, anche se il virus - come auspichiamo - diventasse endemico, questo comunque non eliminerebbe l'impatto l'impatto che avrebbe sulla popolazione, soprattutto fragile. Se c'è una lezione che abbiamo dovuto imparare da questa pandemia, è che dobbiamo anticipare il virus, prevedere che ci possa essere una nuova recrudescenza e prendere per tempo le misure necessarie.

Sappiamo che la prudenza è la virtù dei forti e quanto abbiamo necessità di uscire più forti da questa pandemia. Il collega che mi ha preceduta, il senatore Romagnoli, parlava di un senso del sé che può diventare un senso del noi. un lavoro psicologico con sé stessi per uscire più forti dalla epidemia. Confidiamo quindi nella prudenza dei cittadini, per cui è chiaro che evitare assembramenti eccessivi o anche prestare attenzione a eventuali sintomi legati alla pandemia essere un segnale importante di autogestione e di conforto per le stesse strutture sanitarie. Domenica scorsa abbiamo celebrato la seconda Giornata nazionale del personale sociosanitario.

Teniamo presente - qualche collega l'ha ricordato - che alla crisi pandemica si è aggiunta una crisi legata al conflitto attuale, a cui si aggiungeranno necessariamente restrizioni di tipo energetico. Due grosse difficoltà come queste potrebbero creare seri problemi anche alla tenuta sociale, economica e sanitaria del nostro Paese. Inoltre, è bene ricordare che esiste anche il problema del *long* Covid - ne abbiamo discusso in Commissione sanità - di cui ancora non riusciamo a valutare completamente l'impatto. Conosciamo, però, molte persone che hanno avuto la malattia e presentano ancora dei sintomi, tipo astenia, difficoltà respiratorie cardiovascolari, di cui non conosciamo ancora gli esiti e lo sviluppo. Da parte nostra, da parte della politica, dobbiamo avere una maggiore sorveglianza e prevenzione, soprattutto - per esempio - sul tema dei trasporti. Probabilmente dobbiamo fare ancora molto di più. Siamo molto contenti che la scuola sia tornata in presenza. Siamo una forza politica che ha tanto insistito perché la scuola e l'università potessero tornare in presenza, perché anche in tale ambito i danni psicologici saranno misurati sul lungo termine. Recentemente è stato approvato anche il *bonus* psicologo dall'altro ramo del Parlamento e in questo Camera abbiamo avuto tantissimi emendamenti in Tra qualche giorno saranno trascorsi due anni dal *lockdown*; due anni terribili che hanno cambiato anche le nostre esistenze. Abbiamo perso il gusto della normalità pian piano dobbiamo riprenderlo per uscire da una pandemia che ci ha lasciato anche degli strascichi psicologici. Naturalmente il Governo e il Parlamento in questo periodo hanno dovuto restringere o ampliare le misure a seconda dell'andamento della curva epidemiologica.

Altra lezione della pandemia che non dobbiamo dimenticare è che chi protegge se stesso protegge gli altri: questo è molto importante. È stata quindi una misura necessaria. Nessuno di noi è contento per l'andamento delle conversioni in legge dei decreti-legge, perché anche noi oggi - la giornata lo dimostra - non abbiamo avuto la possibilità di intervenire con un'attività emendativa.

sia nel merito, perché noi vorremmo - come abbiamo chiesto più volte - l'abolizione del *super green pass*, sia perché ci ritroviamo di nuovo all'ennesima richiesta di fiducia da parte del Governo. Fratelli d'Italia è per il no alla fiducia a questo Governo, ma vorrei motivarlo. Siamo contrari perché il Governo ha dimostrato la sua incapacità nella gestione della pandemia, anche perché - dobbiamo dirlo con chiarezza - vediamo che tutti i dati ci confortano da questo punto di vista. Abbiamo visto il calo dei contagi, il calo delle terapie intensive (ormai è nettamente sotto il 10 per cento), il calo dei ricoveri

Dovreste invece prendere atto, anziché della narrazione e del racconto che questa maggioranza fa agli italiani, del fatto che la gestione della pandemia non ha avuto successo. Lo dico con grandissimo dispiacere.

I dati ci dicono che gli italiani sono stati straordinari nel farsi vaccinare, nonostante tutta la confusione, anche dal punto di vista della comunicazione, che questo Governo ha fatto sui vaccini.

creando sicuramente confusione, paura, dubbi e domande da parte degli italiani. Nonostante tutto questo, però, nonostante l'incapacità, da parte del Governo, di gestire anche la comunicazione e l'informazione coi cittadini italiani,

allora, dovrebbe prendere atto che chi voleva vaccinarsi si è vaccinato e chi non l'ha fatto oggi non crediamo possa cambiare idea: magari lo farà una piccola parte, ma non tale da cambiare sostanzialmente i numeri dei vaccinati. Ricordo, anche qui, la confusione fatta dal Governo, dando i dati sulla famosa copertura che dovevamo avere per essere sicuri che il virus circolasse meno tra gli italiani. a oggi questi dati sono completamente scomparsi. Perché, allora, continuare con il *super green pass*? Perché continuare,

Tra i nostri emendamenti, che naturalmente sono stati bocciati, c'era proprio la richiesta dei tamponi salivari. Invece, voi oggi decidete che gli *over* 50 non possono lavorare, non possono quindi ricevere uno stipendio, non possono dare continuità

che sta arrivando in maniera molto pesante, in maniera trasversale, che quindi colpirà tutti. E voi continuate in questa decisione di togliere il lavoro, di togliere lo stipendio ai lavoratori *over* 50. Io sono un po' basita, perché credevo che il sindacato, che in Italia, almeno a parole, si è sempre riempito la bocca con la difesa dei

Fate le cose e poi ne attuate delle altre. Come vi sentite davanti agli italiani quando per voi il tampone va bene oltre i vaccini? Quella mattina io non ho capito perché, fatto tutti e tre i vaccini, dovevo sottopormi al tampone. C'è qualcosa nei vostri fatti e nella vostra narrazione che non torna e guardate che il tempo è galantuomo da questo punto di vista. La verità infatti verrà fuori e sarete smentiti dai fatti.

che non potranno mettere insieme il pranzo con la cena per i loro figli? Nonostante i dati che tutti voi conoscete e che vi ho ricordato, continuate a sbagliare. Fratelli d'Italia non ci può stare e non perché siamo contro i vaccini; voglio dirlo con chiarezza. Non solo parla una persona che ha fatto naturalmente tutte e tre le dosi anche che noi abbiamo sempre detto che i vaccini erano assolutamente fondamentali nella lotta al Coronavirus perché salvavano dal cimitero e dall'ospedale, certamente non dal contagio. Non voglio ricordare nemmeno quando il 22 luglio dell'anno scorso il presidente del Consiglio Draghi in una conferenza stampa disse a tutti gli italiani che il *green pass* dava la sicurezza di frequentare luoghi sicuri *(Applausi)*, perché non era possibile il contagio.

avevamo ragione perché il vaccino non esclude dal contagio. È vero, e lo dico con forza, che esclude la malattia grave.

e poi, molto spesso, le vostre bocche si riempiono di una parola che si chiama democrazia. Signor Presidente, colleghe, colleghi, l'imprevedibile ha fatto irruzione nella nostra vita, prima con una pandemia ed ora con una guerra poco distante da noi. In queste ore tutta la nostra attenzione è rivolta a ciò che sta accadendo al confine orientale del nostro continente, dove la Russia ha deciso di intraprendere un'aggressione violenta contro uno Stato libero e sovrano. Vorrei ribadire la nostra vicinanza ai bambini, alle donne, agli uomini che stanno soffrendo pene indicibili e alle persone bisognose di cura ed assistenza anche in relazione alla loro situazione vaccinale. Ecco, in questo quadro internazionale, così allarmante, continuiamo giustamente a fare il nostro lavoro che in questo caso riguarda l'altra grande emergenza del nostro tempo, la pandemia. Il Governo Draghi ha affrontato la recrudescenza pandemica dei mesi scorsi con provvedimenti fortemente sostenuti dal Partito Democratico e fondati sui principi della gradualità, del rischio ragionato, della prudenza in relazione ai dati scientifici nazionali e internazionali, per cercare di preservare le nostre vite. Una scelta che - dobbiamo dirlo chiaramente - ha pagato, perché, nei mesi difficili tra novembre e gennaio, mentre molti altri Paesi erano costretti a richiudere o a tornare indietro rispetto alle iniziali aperture, noi abbiamo saputo gestire la fase acuta senza assumere misure draconiane che avrebbero ulteriormente penalizzato cittadini, imprese e famiglie. Il Covid, infatti, si combatte non con la propaganda, ma con un approccio serio e progressivo, basato sui dati e non sulle opinioni. La campagna vaccinale - siamo terzi in Europa per dosi somministrate - ci ha consentito di fronteggiare con responsabilità i momenti difficili, ed è per questo che abbiamo sostenuto la necessità di introdurre l'obbligo vaccinale per gli *over* 50. Inoltre, l'estensione dell'obbligo vaccinale anche per il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, degli istituti tecnici superiori; l'estensione dell'impegno delle certificazioni verdi per i servizi alla persona, per gli uffici pubblici, per i servizi postali, bancari, finanziari, per le attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali) sono alcune delle misure che hanno permesso concretamente di contenere i contagi, i ricoveri, i decessi e contestualmente hanno consentito alla nostra economia di ripartire. Le nuove misure annunciate sono volte a permettere una progressiva *road map* in questa direzione, che tiene insieme la tutela della salute e la ripresa economica. Secondo tema degno di attenzione è quello relativo al *green pass*. Conosciamo bene le polemiche strumentali in tanti casi - che hanno riguardato questo strumento. Ebbene, alla Camera sono state introdotte modifiche che vanno lette in relazione al cambiamento del quadro epidemiologico attuale, molto diverso da quello in cui era stato varato il decreto-legge. Tuttavia, mi preme sottolineare che il *green pass* è stato uno strumento importante, che ha incentivato le vaccinazioni e offerto un messaggio chiaro i cittadini che si sono comportati in modo responsabile. Ricordiamoci anche che il Covid ha avuto un effetto devastante indiretto su molti altri ambiti sanitari: gli *screening* oncologici, i trattamenti chemioterapici, la cura delle malattie croniche. Ebbene, i vaccini hanno consentito di ridurre la pressione sugli ospedali e, aumentata la platea dei vaccinati, si è potuto tornare a una gestione clinica che ha rimesso al centro le tante persone sofferenti in questi lunghi mesi. Ancora, l'introduzione del principio di diritto di continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, negli *hospice*; le nuove misure per gestire i casi posti dalle scuole nelle competizioni sportive e l'introduzione del principio del diritto di continuità sono i tantissimi nuovi elementi che danno il senso di serietà alla strada percorsa.

In questo senso, sono felice del lavoro che sta portando avanti il Partito Democratico e qui, al Senato, il nostro Gruppo. Segnalo in particolare due questioni: anzitutto è importante aver stabilito che le istituzioni scolastiche siano in ogni caso tenute a garantire e a rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione e di riorganizzazione delle attività. La seconda è un segnale molto forte e importante, l'istituzione del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione, attraverso attività gratuite extrascolastiche, attività culturali, sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio, sostegno psicologico e pedagogico. Il Covid-19 ha profondamente cambiato il volto della nostra comunità, rimettendo in primo piano

era e rimane un elemento fondamentale di ricostruzione e di sviluppo di comunità, perché è l'istituzione indispensabile per tenerla unita, farla crescere e permettere ai più giovani di partecipare, di essere inclusi nella vita collettiva. Purtroppo la pandemia ha allargato le differenze e ha fatto emergere nuove fragilità nel tessuto sociale. Soprattutto i ragazzi hanno risentito degli effetti delle restrizioni, a partire dalla mancanza della didattica in presenza, che ha aumentato le disuguaglianze nei percorsi educativi, nelle possibilità di apprendimento e in quelle relazionali. Ricordiamo che ci sono 10 milioni di cittadini *under* 18 che non hanno alcuna forma di sostegno, salvo il lavoro eccellente delle organizzazioni del terzo settore. Ora la sfida nei prossimi mesi sarà proprio quella di rafforzare e ricostruire le alleanze educative, di allargare le reti di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e il terzo settore, con tutte le associazioni che operano sul territorio, dai centri sportivi agli oratori. Questo è lo strumento per potenziare l'offerta educativa dalla più tenera età fino a quella adulta: sostenere le famiglie, combattere la dispersione scolastica e la povertà minorile, ricucire il tessuto sociale rimettendo al centro la persona e la crescita. L'incrocio di tutti questi mondi dovrebbe gravitare intorno alla scuola, costruendo dei patti educativi di comunità basati su due elementi indissolubili: la co-progettazione e la co-responsabilità dell'azione educativa. Dobbiamo trovare le strade per tornare verso i più giovani, co-costruire comunità per ripartire insieme. Nel frattempo è urgente proseguire con la gradualità e la razionalità che hanno caratterizzato l'azione del Governo, perché la tempesta non è alle spalle e serve lungimiranza e visione. Il Paese ha bisogno di costruire il proprio futuro e non di una campagna elettorale permanente. Mi auguro che tutte le forze politiche dimostrino fermezza e responsabilità in questa direzione. Signor Presidente, colleghi, colleghe, Governo, oggi possiamo dire che la grande paura l'abbiamo lasciata alle spalle. La linea della prudenza e della gradualità sembra aver pagato. I giorni delle file chilometriche per i tamponi davanti alle farmacie, delle sirene delle ambulanze per gli ospedali, delle polemiche e delle manifestazioni di chi testardamente aveva deciso di non vaccinarsi sembrano lontani, anche perché in queste ore siamo tutti rivolti a un'altra emergenza drammatica, che mette in discussione la democrazia e la libertà nella nostra Europa. Ci troviamo a fronteggiare una guerra che è dentro i confini della nostra Europa; dovremmo dire "vicino" più che "dentro", ma nel nostro Paese vivono già decine di migliaia di donne e uomini ucraini a cui va la nostra solidarietà. Non li lasceremo soli a combattere la Russia di Putin che ha invaso il loro Paese. Oggi siamo in Aula per esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio scorso, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Diciamoci la verità: tutti noi contiamo i giorni che mancano al 31 marzo, all'annunciata fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid. Solo due mesi fa c'erano più di 108.000 contagi al giorno, che ieri si sono più che dimezzati (46.631); certo, i decessi sono ancora troppi (233), ma i dati che fanno ben sperare sono il tasso di positività, che è sceso all'8,8 per cento, e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive e nelle aree mediche, che con costanza diminuiscono giorno dopo giorno: due mesi fa erano 14.600 i posti letto occupati nelle aree mediche, oggi sono 10.000; due mesi fa erano 1.500 i posti occupati nelle terapie intensive, oggi meno della metà (709). Il bilancio di questi due anni di pandemia è drammatico: 155.000 morti, quasi 13 milioni di contagiati. Però siamo ottimisti - e soprattutto lo è la scienza scienza - perché la campagna di vaccinazione ha funzionato e il vaccino ha salvato migliaia di vite umane. L'83,4 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario,

Questo che ci apprestiamo a votare è il decreto-legge che introduce fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, esclusi ovviamente i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che

generato cioè esclusivamente da vaccinazione o da guarigione per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico e privato e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Ho ascoltato la collega Santanchè, che accusa la Sinistra e i sindacati di non aver difeso i lavoratori. Eppure, proprio la linea del rigore, proprio il *green pass,* proprio i vaccini hanno consentito a questo Paese di continuare a marciare, hanno salvato le aziende, la nostra economia e quindi i lavoratori. Per questo non capisco questa sottolineatura della collega Santanchè. Sappiamo bene che è stata una misura dolorosa e tutti ci auguriamo che, con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo, si possano progressivamente eliminare molte limitazioni che questo comporta. Dico al Governo che io mi auguro che possa cessare il *green pass* rafforzato nei luoghi di lavoro. Tuttavia, bisogna essere chiari su un punto: fino a quando non lo dirà la scienza, la fine dello stato di emergenza non decreta di per sé la fine della pandemia; di certo si rivedranno i luoghi dove sarà necessario il *green pass,* ma anche oggi l'uscita dagli obblighi dovrà avvenire con gradualità. Non credo che sia già arrivato il momento di convivere con la malattia; certamente non è più necessario indossare la mascherina all'aperto, se non in caso di assembramento, ma al chiuso? Tra otto giorni, in esame, sarà consentito per esempio il consumo di cibi e bevande a teatro, nelle sale da concerto, al cinema, negli stadi che via via si stanno riempiendo. Tutti noi vorremmo evitare queste misure. Tutti noi amiamo la libertà. Non è che chi sostiene o ha sostenuto la linea del rigore non ami la libertà. Tutti amiamo la libertà e tutti pensiamo che la salute di tutti sia stata la nostra ancora di salvezza, scritta nella Costituzione. Gli effetti della variante Omicron, contagiosissima, sono stati fronteggiati perché hanno funzionato vaccini e rigore. Ora possiamo guardare al futuro con più ottimismo, anche se i venti di guerra che soffiano sulla nostra Europa ci preoccupano tantissimo. Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali, vorrei sottolineare due punti, che pongo sempre all'attenzione dell'Aula nei miei interventi. È giunto il momento di riflettere insieme sulla necessità di procedere a una riforma della sanità. Se abbiamo retto, anche se con un bilancio drammatico di vittime, è perché abbiamo potuto contare sulla sanità pubblica, nonostante i tagli e la penalizzazione della medicina territoriale. medicina territoriale. Oggi, che stiamo uscendo dall'emergenza, dobbiamo sforzarci di dare organicità e di affrontare i nodi non risolti, per fare un salto di qualità. per tornare alla vita normale, dobbiamo mettere in sicurezza il pianeta e vaccinare tutti, anche le donne e gli uomini che vivono nei Paesi poveri, perché il Covid non conosce frontiere. Dunque votiamo "sì" alla fiducia come senatori di LeU-Ecosolidali.

Ho ascoltato con attenzione il dibattito e ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi delle altre forze politiche. Devo dire da questo punto di vista che a volte, proprio perché

via via accaduto e le tante sterzate e richieste a cui abbiamo assistito. Una volta si protestava perché si doveva aprire; poi si protestava perché si doveva chiudere; poi si protestava perché le scuole erano aperte; poi si protestava perché erano chiuse; poi si protestava per il vaccino; poi si protestava perché magari non c'era l'obbligo per i medici. Insomma, io credo che il punto fondamentale

di un percorso, che è stato seguito da un anno a questa parte con la precisa volontà di tenere la barra dritta su determinate questioni.

e soprattutto abbiamo una prospettiva molto chiara con riferimento alla fine dello stato d'emergenza. I colleghi, nei loro precedenti interventi,

Sono stati approvati degli emendamenti, con riferimento in modo particolare all'assistenza delle persone con problemi di capacità cognitiva

siamo talmente scossi da quello che è accaduto in Ucraina che a volte, nel parlare di pandemia, ci sembra di affrontare un problema più piccolo, rispetto a uno molto più grande.

quello che è successo e sta succedendo in Ucraina ci faccia capire che le parole vanno pesate. Quando si parla di libertà e

una dittatura, e comunque una situazione di violazione delle libertà. Possono esserci delle limitazioni per il rispetto e soprattutto per la tutela di altri diritti e ci possono essere invece delle violazioni che sono un sopruso e una vera dittatura.

Tra l'altro, questo provvedimento oggi diventa un po' anacronistico, perché due mesi fa poteva avere le sue giustificazioni sulla base dei dati molto allarmanti

che non sono vaccinati finiscano in DAD rispetto a chi è vaccinato. Questa è una discriminazione, anzi - parliamoci chiaro - è un obbligo mascherato che noi non abbiamo condiviso, innanzitutto perché stiamo parlando di bambini. *(Applausi).* Tra l'altro, qualcuno - lo dico al sottosegretario Sileri - ci deve spiegare perché c'è tutta questa insistenza sui bambini dai cinque agli undici anni solo in Italia,

C'è anche un altro tema che è stato introdotto in questo decreto con un emendamento: la differenza di trattamento tra gli italiani e gli stranieri. Se uno straniero arriva in Italia ha fatto due dosi di vaccino da più di sei mesi, basta il tampone e può benissimo entrare in albergo o andare al ristorante. Il cittadino

ci mancherebbe altro - noi abbiamo il Ministro del turismo e siamo i primi a essere soddisfatti da questo punto di vista - ma non possiamo fare una discriminazione tra un cittadino europeo e un cittadino italiano.

*green pass* diventa uno strumento politico e non più uno strumento sanitario. Se non siamo in emergenza, che ragione c'è di mantenere il *super green pass*, il *green pass* e altro? Anzi, sono gli stessi virologi che consigliano, visto che la situazione in questo momento è molto migliorata e si presume che a fine marzo sarà ancora migliore, dare libertà ai cittadini, visto che non sappiamo a ottobre che cosa potrebbe capitare. Ci auguriamo che vada tutto bene e che la pandemia sia finita, possiamo pensare eventualmente a delle restrizioni se le cose dovessero non andare bene nel periodo autunnale. È questo il periodo in cui garantire libertà e serenità a tutta la popolazione. È adesso il momento di farlo e non arrivare fino a giugno.

già adesso con lo stato d'emergenza delle sentenze del TAR del Lazio hanno sospeso il provvedimento di mancato stipendio a coloro che non vogliono vaccinarsi, perché i giudici ritengono necessario un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della salute e il diritto al sostentamento. In questa fase, con l'arrivo addirittura della guerra, con tutte le difficoltà economiche e l'aumento delle bollette,

Signor Sottosegretario, tutti qui la pensano alla stessa maniera; quasi tutti. Non abusate della pazienza dei cittadini e del Parlamento, perché c'è un'unità di consensi. Dal 1° aprile arriverà qualche provvedimento in Aula e ci sarà qualche votazione dell'Assemblea. Quindi ditelo al ministro Speranza, tra l'altro fondatore del partito che si chiama Articolo Uno. L'articolo 1 della Costituzione

Ricordateglielo, con eleganza e in modo garbato, perché conosciamo il suo carattere. Quindi, ci mancherebbe altro, usate tutte le precauzioni, ma ricordateglielo, visto che è tuttora segretario di quel partito. Ho parlato dei

in un momento particolare di difficoltà, di fase acuta della pandemia, ci sta che ci siano dei provvedimenti restrittivi. Ma se le cose vanno meglio e tutti pensiamo giustamente che dobbiamo combattere per difendere la democrazia e la libertà, cominciamo a difendere la libertà dei nostri connazionali.

Il risultato qual è? Il grido d'allarme delle associazioni oncologiche italiane, con gli *screening* che sono stati quasi tutti bloccati.

approvata dal Parlamento il 22 dicembre 2017, prevedeva di apportare notevoli benefici alla ricerca sui tumori pediatrici. Tutt'ora, signori Sottosegretari e signori Ministri, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. Com'è possibile? Giusta la battaglia, giusto tutto l'impegno. Io ringrazio il Ministero per tutto quanto è stato fatto nella lotta al Covid-19 e per tutto quello che continuate a fare. Colleghi, non esiste, però, solo il Covid-19. Si muore per tante altre patologie e sono tanti i bambini che avrebbero bisogno di quei decreti attuativi.

che oggi l'Assemblea sta discutendo e che approverà, non si può non considerare il fattore temporale, cioè la collocazione nel momento esatto in cui esso è stato programmato e deciso dal Governo. Ovviamente, in quel momento la situazione epidemiologica della pandemia - come già ribadito da molti - le curve dei contagi e i tassi di occupazione delle nostre terapie intensive e dei posti letto Covid-19 nelle strutture ospedaliere davano, nell'insieme, segnali molto preoccupanti ed estremamente differenti da quelli attuali. Essi, nell'insieme, non lasciavano intravedere quel graduale e progressivo miglioramento della situazione generale che, al momento attuale, ci pone in uno stato di relativa tranquillità

dall'altro, di guardare con fiducia al futuro e alla fine dello stato di emergenza, previsto per il 31 marzo 2022. Dalla valutazione oggettiva dei dati rilevati e della realtà epidemiologica nelle diverse ondate epidemiche, nelle fasi di acutizzazione e nelle risalite dei contagi non si può non riconoscere il ruolo fondamentale svolto, in senso estremamente positivo, dal progredire della campagna vaccinale. I diversi provvedimenti adottati, pur con le ovvie e oggettive difficoltà generali, collegate alla situazione economica, sociale e sanitaria del nostro Paese, hanno seguito una logicità e un percorso fondato sui dati scientifici e sui suggerimenti della cabina di regia, dopo aver fatto le opportune valutazioni politiche. La stessa adozione del *green pass* è stato sia uno strumento di protezione, per i soggetti vaccinati, sia - al tempo stesso - un mezzo per tutelare coloro che non si sono vaccinati, gli esitanti e i riottosi. L'adesione responsabile alla campagna vaccinale sicuramente ha ricevuto un notevole impulso dall'adozione di questa misura. Voglio credere che le campagne informatrici e di sensibilizzazione, sempre più capillari e soprattutto capaci di motivare, abbiano spazzato via molte delle perplessità e delle titubanze dei tanti incerti e restii a vaccinarsi; quasi che le tante decine di migliaia di vite spezzate dalla violenza e dalla aggressività del virus fossero solo un cattivo sogno o quasi una situazione surreale. Al contrario esse sono state e costituiscono tuttora una tristissima e cruda realtà. L'obbligo del *green pass* ha dato senza dubbio una spinta importante alla campagna vaccinale permettendo di reclutare i cittadini indecisi e non recettivi alle indicazioni scientifiche. L'importante era raggiungere la percentuale più ampia possibile di vaccinati e ciò è stato fatto. fatto. Attualmente circa il 90 per cento dei soggetti ha completato il ciclo vaccinale e ci stiamo avviando verso l'immunità di gregge o di comunità. Questi dati pongono il nostro Paese ai primi posti nel mondo per percentuale di popolazione vaccinata. In quest'ottica la misura dell'obbligo vaccinale per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, norma prevista in questo decreto-legge, con le ovvie esclusioni in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi che comprendono i soggetti in cui sussistono controindicazioni cliniche alla vaccinazione e per quelli che hanno contratto precedentemente il Covid-19, vuol essere un ulteriore mezzo per proteggere quelle fasce di età secondo dati statistici evidenti ed oggettivi, gli effetti deleteri della virulenza e della patologia da Covid sono molto più gravi, progressivi e, a volte, inarrestabili. La rapida progressione della malattia si osserva essenzialmente nei non vaccinati o quando sussistono condizioni patologiche concomitanti più o meno conosciute. I dati riportati sulle percentuali dei posti occupati nelle terapie intensive Covid dedicate fotografano con chiarezza la realtà e sono incontestabili, con un rapporto dell'80 per cento circa dei soggetti non vaccinati e del 20 circa di quelli vaccinati (questi ultimi sempre con patologie gravi concomitanti). Vorrei inoltre ricordare che le forme sintomatiche sono capaci di far sentire le loro ripercussioni cliniche sulla qualità della vita dei pazienti anche negli anni successivi con la sindrome *long* Covid, entità patologica riconosciuta e sempre più frequente. Come tutti sappiamo, a fine marzo terminerà lo stato d'emergenza, come ha già sottolineato il presidente Draghi. Come ha ribadito anche il nostro presidente Conte, questo risultato è il frutto degli sforzi e della resilienza di tutti i cittadini e della nostra collettività. Abbiamo attraversato momenti difficili, con un percorso di grande sofferenza; ora guardiamo al futuro con fiducia e alla prospettiva di un ritorno alla normalità. Occorre avviare un piano per allentare gradualmente tutte le misure, un piano complessivo di revisione dei provvedimenti anti-Covid, alla luce - come già detto - del miglioramento della curva epidemiologica e dell'alleggerimento della pressione sulle strutture sanitarie. Se siamo arrivati a questo punto, non si può comunque non riconoscere l'efficacia delle misure adottate. In questa nuova fase occorrono modifiche e iniziative che contemplino il giusto bilanciamento del diritto alla salute con il diritto al lavoro, consentendo un'efficace e decisa ripartenza economica insieme a un graduale ritorno alla vita sociale e culturale. Non abbiamo bisogno però di brusche accelerazioni, che potrebbero successivamente comportare altrettante rapide frenate. Si deve attuare una progressione graduale, che - da un lato - guardi, alle giuste richieste delle attività imprenditoriali, commerciali, economiche e produttive del nostro Paese e, in generale, alle necessità di socialità sollecitate da tutti i cittadini, ma che - dall'altro - tenga sempre conto dei suggerimenti della scienza e delle valutazioni della realtà epidemiologica nel suo stato attuale e nella prospettiva futura. In quest'ottica va la richiesta di un confronto globale da parte del presidente Conte e di tutto il MoVimento 5 Stelle, che comprenda anche la revisione del *green* *pass*, con un piano graduale per l'eliminazione del suo utilizzo. Non si tratta di essere più o meno aperturisti o di far passare il messaggio - sbagliato, secondo me - del liberi tutti; occorre essere semplicemente realisti ed equilibrati. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre mostrato, nella gestione pur difficile e, a volte, controversa della pandemia, coerenza, senso di responsabilità, lealtà e impegno, nel solo interesse dei cittadini. Pertanto, anche a questo provvedimento darà il suo voto favorevole. *(Applausi).*

ed evidentemente il ricatto è lo stesso che stanno subendo gli italiani che, se non si vaccinano, non possono andare a lavorare; e, se non lavorano, non hanno uno stipendio. Domando allora al Governo: ma come devono campare gli italiani?

pessima, ingannevole e ipocrita questione burocratica. Ecco perché gli italiani ormai hanno aperto gli occhi e stanno perdendo la pazienza. Qualcuno pensa che tanto gli italiani dimenticheranno. No,

stipendio per portare avanti una battaglia di resistenza che ha tutto il sacrosanto diritto di essere rispettata. E voi non lo state facendo, perché ancora una volta ponete una questione di fiducia

pieno di tensioni? Hanno vissuto anche gli scontri degli adulti: almeno un po' di palestra fategliela fare, senza obbligatorietà di questo *green pass*! di altre questioni che ormai sfuggono completamente a qualunque logica? Non abbiamo più un nome e un cognome: siamo un quadrato magico; quante volte abbiamo dovuto dovuto dimostrare di essere qualcuno, di essere titolari di un diritto mostrando un quadrato magico? Neanche la carta d'identità viene mostrata con tanta frequenza. Direi di finirla. Avevamo la possibilità di resettare tutto prima con la questione pregiudiziale - ma avete detto di no, con il voto direte di no, perché c'è la fiducia nei confronti di un Governo che compie soltanto ricatti. Cari parlamentari, cari colleghi, allora sta a voi l'ultima decisione, ma gli italiani non dimenticheranno.

in questi anni. Eppure quello che, in definitiva, è un provvedimento politico ha ricadute anche su quest'Assemblea, oltre che sul lavoro. Si tratta perché, per un provvedimento politico e non sanitario, in quest'Aula è arbitrariamente impedito ad alcuni rappresentanti eletti dal popolo di essere presenti e di votare, qui e oggi. pregiudizio grave, che oggi - direte - non fa la differenza, ma che, in linea di principio e senza pregiudizio di valutazione, la potrebbe fare, se non ci fosse l'evidente

votando la conversione di questo decreto-legge proseguite su una strada di imposizioni, di obblighi, di burocrazia e di vessazioni che non hanno niente a che vedere con le necessità sanitarie, quanto meno di questo momento. Eppure, da tanti colleghi

di fronte a questo, non bastano i distinguo. Questa è una cosa che rimarrà gli atti: si vedrà chi ha votato a favore e chi ha votato contro. Il tempo è galantuomo e ci si ricorderà in futuro di quello che state facendo. Adesso avete l'ultima occasione per riprendervi, perché fino adesso avete votato tutte le follie che vi ha detto questo Governo. Questo è l'ultimo momento utile: ricordatevelo.

n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: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 Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo.

approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Signor Presidente, siamo qui oggi per approvare in quarta lettura il testo delle disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il testo che avete nelle vostre mani è fortemente atteso dal mondo dell'agricoltura in generale e dell'agricoltura biologica in particolare, proprio perché fornisce tutta una serie di strumenti fondamentali per affrontare le sfide che l'agricoltura in generale e l'agricoltura biologica in particolare hanno di fronte, soprattutto alla luce degli obiettivi della nuova Politica agricola comunitaria e

che - come dicevo - è molto atteso dal mondo agricolo, affronta e mette in campo tutta una serie di strumenti, che partono da un tavolo tecnico di programmazione che ha l'obiettivo di attivare un piano d'azione nazionale per la conversione al biologico,

prevede la definizione di un marchio dell'agricoltura biologica realizzata nel nostro Paese; questo è particolarmente importante, proprio perché in Italia l'agricoltura biologica è oggetto di grande attenzione, di controllo, di verifica e di certificazione, cosa che non avviene in tutta Europa e in tutto il mondo. Poter dire che un certo prodotto è stato realizzato con i canoni, i controlli e le verifiche della nostra agricoltura è uno strumento assolutamente fondamentale per i consumatori. Viene messo in campo un piano nazionale per le sementi, viene attivato un fondo di sviluppo per l'agricoltura biologica, vengono sostenuti le integrazioni di filiera, la ricerca di settore, di settore, i percorsi di formazione professionale, i distretti del biologico, la disciplina delle organizzazioni interprofessionali e quella delle organizzazioni di prodotto. Vengono sostenuti gli accordi quadro e le intese di filiera, viene definito in modo giuridicamente puntuale tutto il tema della certificazione delle sementi e viene data la delega al Governo per una revisione, un'armonizzazione e una razionalizzazione delle norme sui controlli. Questo è il tema del disegno di legge al nostro esame.

21, l'azione delle clausole di salvaguardia, che non agiscono più soltanto sull'attuazione della norma, ma anche sull'attuazione dei decreti legislativi

producesse una legge degna di questo nome, per disciplinare il marchio. Il mercato del biologico, secondo Nomisma, nel 2020 aveva raggiunto i 6,9 miliardi di euro,

Devo dire che sono molto rattristata dal fatto che il disegno di legge in esame abbia avuto un *iter* così lungo, perché si è voluto sin dall'inizio introdurre al suo interno la pratica dell'agricoltura biodinamica

Stavo dicendo che sono molto rattristata dal fatto che l'*iter* del disegno di legge sia stato rallentato dall'aver voluto introdurre sin dalla prima lettura il termine «biodinamico» all'interno del disegno di legge. È stato questo a rallentare l'*iter*; è stato questo il motivo per cui oggi ci ritroviamo alla quarta lettura, altrimenti avremmo dato questa opportunità ai nostri

che tra l'altro grava chi lo richiede di costi aggiuntivi. Voglio portare la voce degli agricoltori, che in questo momento soffrono molto, sia per la pandemia, sia per lo sconvolgimento internazionale. L'emergenza attuale è garantire agli agricoltori un prezzo equo per i prodotti agricoli. La Commissione agricoltura si sta occupando da tempo del disegno di legge sul prezzo minimo garantito agli agricoltori e invito quest'Assemblea a considerare che tutti noi, al di là delle chiacchiere, ci nutriamo poi di cibo vero, quello che producono gli agricoltori. Il rischio è che non ce la facciano più a portare il cibo sulle nostre tavole, se continuiamo ad approvare leggi

Dobbiamo finirla di guardare all'agricoltura come al mondo dei delfini, dei papaveri e delle viole, come spesso si dice, perché è un mondo nel quale ci sono degli imprenditori seri e preparati, che sostengono la nostra economia e il nostro il nostro Paese, portando sulle nostre tavole l'agroalimentare migliore del mondo. Ci vuole dignità e ci vuole la considerazione di questo settore come un settore imprenditoriale importante e difficile.

Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, finalmente oggi siamo qui a votare definitivamente questo provvedimento che, parlando di imprenditori agricoli e di agricoltori, tanto atteso nell'ambito dei lavori parlamentari. In questo periodo difficile in cui nella fase *post*-pandemia e nell'attuale fase bellica l'economia è in difficoltà, c'è bisogno di risposte. L'agroalimentare italiano è una pietra miliare della nostra economia va sostenuto. Esso sarà il traino futuro dell'economia; ci sarà bisogno di beni, ma, soprattutto di prodotti sani e genuini, che possano essere utilizzati per fare appunto da traino a tutta l'economia. All'articolo 1 viene definita la produzione biologica quale sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basata sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente, azione per il clima e salvaguardia delle risorse naturali.

così come produrre biologico: è una scelta di principio, ma anche un'opportunità economica, vista la richiesta dei consumatori, sia in Italia che nel mondo. Non diventi, però, l'agricoltura biologica, l'antitesi dell'agricoltura con metodi convenzionali: sono due realtà che possono e devono coesistere. Tornando al testo del provvedimento, l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, contraddistinti dall'indicazione "biologico italiano", che è una tutela per gli agricoltori e per i produttori ed una garanzia per i consumatori, visto che certificherà prodotti biologici realizzati con materie prime al 100 per Al di là delle polemiche che sono nate anche in questi giorni, il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare chiede risposte subito. È un segnale, in un provvedimento tanto atteso, non bisogna tergiversare perché è grazie a questo provvedimento che l'economia agricola e agroalimentare trarrà maggiori benefici

intervengo in questa discussione generale perché vorrei ripercorrere con voi alcuni passaggi di questo disegno di legge che credo importanti e positivi e vorrei, con questo, anche anticipare a voi la presentazione di un ordine del giorno che poi verrà rimesso all'Assemblea. Vorrei partire dallo scorso 20 maggio, quando in quest'Aula presentai tre emendamenti sulla legge oggi in discussione, volti ad eliminare i riferimenti espliciti all'agricoltura biodinamica, soprattutto per quanto riguarda la sua equiparazione all'agricoltura biologica, al comma 3 dell'articolo 1. Devo dire che mi sentii in dovere, in quella giornata, di leggere in Aula una parte delle pratiche esoteriche che fanno parte dell'agricoltura biodinamica e mi ricordo che molti tra voi colleghi mi hanno riferito che quando il disegno di legge è arrivato in votazione non sapevano esattamente cosa fosse la biodinamica dopo averlo appreso, alcuni di voi mi hanno riferito di essersi chiesti come sia stato possibile menzionare certe pratiche nel testo finale di una legge dello Stato nel 2021, mentre la scienza veniva, come viene tutt'ora, esaltata da tutte le parti per il suo ruolo nel combattere la pandemia. Vi ricordo che quei tre emendamenti hanno raccolto fra i 30 e i 40 voti favorevoli, ma la grande maggioranza dei senatori aveva scelto di bocciarli, molti anche - mi è stato poi spiegato - con la motivazione di non rallentare l'*iter* della legge. L'unico voto contrario in Aula fu il mio, l'unica astensione quella della senatrice Fattori e il testo è tornato alla Camera. In Commissione agricoltura, nel luglio dello scorso anno, la maggioranza dei deputati, sempre per non rallentare l'*iter* della legge, ha rigettato qualunque emendamento su questo argomento e questo - e mi rincresce - nonostante molte società scientifiche si fossero coordinate in una mobilitazione senza precedenti per aiutarci contro il rischio di legittimare il pensiero magico in una norma di rango primario di iniziativa del nostro Parlamento. Sei tra le maggiori società scientifiche italiane del settore agricolo

che raggruppano i nostri esperti e i nostri studiosi. Le voglio ricordare: l'Associazione italiana società scientifiche agrarie, l'Accademia nazionale dell'agricoltura, la Federazione italiana scienze della vita, l'Unione nazionale delle accademie per le scienze agrarie, l'Accademia nazionale delle scienze, l'Accademia dei Georgofili. Accanto alle società già citate si sono mobilitate molte delle più autorevoli istituzioni scientifiche e di ricerca italiane: mi riferisco all'Accademia dei Lincei (anche organo di consulenza scientifica della Presidenza della Repubblica), alla Società italiana di tossicologia, alla Società italiana di genetica agraria, alla Conferenza dei rettori delle università italiane. Ebbene, dopo uno *stop* di più di sei mesi, l'8 febbraio scorso il disegno di legge è approdato in Aula alla Camera e nell'ultimo momento utile i deputati, con 421 voti favorevoli e nessun contrario, hanno deciso di intervenire in maniera netta e inequivocabile per rimuovere da un disegno di legge in via di approvazione il riconoscimento di pratiche esoteriche e ascientifiche. A quanto ho appreso, la decisione della Camera è stata frutto della volontà di far tesoro anche delle rassicurazioni che il presidente Mattarella aveva indirizzato al professor Giorgio Parisi, Nobel per la fisica, lo scorso novembre inaugurando l'anno accademico della Sapienza di Roma. Il professor Parisi, già dall'estate precedente, quando era presidente dei Lincei, aveva sollevato la ferma preoccupazione relativa alla presenza di riferimenti espliciti alla biodinamica nel disegno di legge in via di approvazione, da lui definita «una pratica francamente stregonesca». Desidero menzionare, proprio in relazione all'attività della Camera, in particolare l'onorevole Riccardo Magi che, sia in Commissione che in Aula, ha presentato e difeso emendamenti volti a sopprimere quell'equiparazione tra biologico e biodinamico. Credo non si possa non ringraziare tutta la Commissione agricoltura della Camera nella sua interezza, il Governo tutto, a partire dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, oltre ai 421 deputati. Credo che solo grazie a questo impegno corale quell'equiparazione è stata eliminata dall'oggetto e dalle finalità dell'articolo 1 del suddetto provvedimento. Che ci fossero problemi ordinamentali, del resto lo aveva rilevato anche il Comitato per la legislazione in un parere che invitava la Commissione della Camera a riconsiderare l'equiparazione tra biologico e biodinamico poiché di quest'ultimo non esiste una definizione legislativa. Da parte sua, l'Ufficio legislazione straniera della Camera ai primi di giugno dell'anno scorso segnalava come l'agricoltura biodinamica, pur liberamente praticata, fosse assente da ogni richiamo nella legislazione di Francia, Spagna e persino Germania, sede di Demeter international, la multinazionale della certificazione biodinamica. Eppure, nonostante l'accordo di tutti i Gruppi sull'articolo 1, sappiamo che alla Camera non sono stati toccati gli articoli 5 e 8, nel rispetto del principio della doppia conforme. Si tratta di articoli che, pure in forme diverse, promuovono la biodinamica. All'articolo 5 si prevede un rappresentante delle associazioni biodinamiche, ulteriore e autonomo rispetto a quelli dell'agricoltura biologica, al tavolo tecnico ministeriale istituito *ad hoc*. All'articolo 8, che disciplina il piano nazionale delle sementi biologiche, c'è il riferimento alle sementi biodinamiche. Colleghi, queste disposizioni oggi appaiono poco comprensibili, visto che è caduta l'equiparazione all'articolo 1 e quindi non c'è ragione di considerare l'agricoltura biodinamica agli occhi della legge come autonoma rispetto all'agricoltura con metodo biologico, che la comprende. Scorrendo il resoconto della Commissione agricoltura del Senato, di mercoledì scorso, ho visto che infatti i colleghi di vari Gruppi avevano sollevato tale questione. La risoluzione di questo aspetto è stata demandata alla presentazione di un ordine del giorno: una modalità su cui hanno concordato molti degli intervenuti in quella discussione. È per questo motivo che ho deciso di presentare in Aula un ordine del giorno aperto alla sottoscrizione di tutti i colleghi che vorranno farlo, e già sottoscritta dai colleghi Zanda, Rizzotti, Fattori, Binetti, Lonardo, Unterberger, Bonino, Richetti, Masini, Quarto, Abate, Bressa, Steger, Laniece, Di Marzio, Durnwalder e Perosino. Questo ordine del giorno ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge sulla revisione del sistema dei controlli e, contestualmente, a sostenere e, contestualmente, sostenere tutte le iniziative legislative volte alla eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con "metodo biodinamico" di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge. di legge. Anch'io vorrei condividere con voi una riflessione sul mondo agricolo, un mondo alquanto complesso, che racchiude una categoria importante di professionisti ed imprenditori, che fanno i salti mortali, veramente, per ottemperare a vincoli che spesso confliggono con le stesse scelte imprenditoriali e che mirano produrre per noi cibo sano e sicuro; una categoria attenta, che deve essere attenta, alla sostenibilità ambientale e a quella economico-sociale. Ogni misura deve essere per questo calibrata, tenendo conto delle evidenze scientifiche disponibili, per dare rilevanza a un principio che va al di là di specifici metodi, cioè quello dell'agricoltura integrata. Una Una concezione laica e scientificamente fondata della sostenibilità, che ci permetta, come italiani ed europei, di non gettare alle ortiche, letteralmente, secoli di eccellenza nel campo della produzione agricola e di dipendere meno dall'estero per il nostro sostentamento quotidiano. Questo è quanto andrebbe comunicato ai cittadini, per incoraggiarli a introdurre più frutta e verdura sulle loro tavole, seguendo le linee guida della sana alimentazione, senza paure infondate, senza bisogno di spendere di più. Questo è l'interesse nazionale che vorrei vedere tutelato da una politica basata sulle evidenze scientifiche. signori del Governo, colleghi, rafforzamento della filiera biologica, marchio biologico unico italiano, distretti biologici, controlli, monitoraggi, analisi dei dati e tracciabilità: questi i temi per noi fondamentali del disegno di legge n. 988, su cui, insieme ai colleghi della Commissione agricoltura di Camera e Senato, abbiamo lavorato negli scorsi mesi siamo felici, oggi, di approvare in via definitiva. Un testo, questo, tanto atteso dai produttori e dalle organizzazioni. Ringrazio il Governo e il sottosegretario Battistoni, per la sua presenza, ma anche per essere un importante punto di riferimento, non solo per noi di Forza Italia. Il comparto agricolo non può non essere sotto i riflettori. Se nel passato questo è successo, dobbiamo oggi, ancor di più, dimostrare il cambio di passo. è sotto i riflettori per gli ottimi risultati economici, essendo tra i pochi in crescita anche durante la pandemia. Penso, appunto, al biologico, che ha registrato una crescita del 5 per cento, con 2,1 milioni di ettari coltivati con metodo bio. Così come per la sostenibilità, dove l'attenzione dei nostri agricoltori nei riguardi dell'ambiente è cresciuta del 57 per cento, ma anche per ciò che il comparto agricolo ha rappresentato e rappresenta in un periodo come quello che stiamo vivendo: certezza del cibo sano sulle nostre tavole. Quindi, è evidente come questa legge fosse prioritaria e di urgente approvazione, ricordando a me stessa che, in Senato, era già stata licenziata a maggio del 2021, in quanto segnale di ascolto di un intero comparto, che da tempo sostiene il nostro prodotto interno lordo, nonostante le innumerevoli difficoltà legate, ad esempio, ai cambiamenti climatici, alle difficoltà di accesso al credito, al reddito degli imprenditori agricoli, sempre più eroso e che, conseguentemente, non rende sostenibili tutti gli investimenti necessari. sostanzialmente note da tempo a chi si occupa di agricoltura, su cui si cerca di lavorare, si sono aggiunte in questi mesi altre allarmanti variabili. Ad esempio il caro energia, che si riflette necessariamente sui prezzi finali e che ha mandato in *tilt* molte aziende: un aumento in termini percentuali insostenibile. Collegato al problema del caro energia c'è poi un altro tragico problema: la guerra in Ucraina. Il mio personale pensiero va al popolo ucraino e alle famiglie di chi purtroppo ha perso la vita in questi giorni. *(Applausi)*. Ciò ha evidenziato ulteriormente la nostra eccessiva dipendenza dall'estero per quel che riguarda il gas e le materie prime. Naturalmente questa guerra si rifletterà sulle scelte dei nostri produttori e sulle tasche dei consumatori con i prezzi di beni essenziali che subiranno ulteriori aumenti nonché diminuzioni nelle produzioni. In questo contesto, la produzione bio, con i suoi disciplinari attenti non solo l'ambiente, ma al consumo di materie prime, alle fonti energetiche, al ridotto consumo di concimi e prodotti fitosanitari, i cui prezzi sono schizzati alle stelle, può e deve rappresentare uno degli alleati alla riduzione delle problematiche elencate. È il caso di dire che il biologico italiano è avanti; lo è in termini di ettari, due milioni in Italia, circa il 16 per cento della superficie agricola utilizzata; lo è rispetto alla media europea di coltivati a bio. La media europea è infatti all'8 per cento contro il 16 per cento italiano. Ricordo che l'obiettivo della comunità europea è l'incremento del biologico al 25 per cento entro il 2050. Dal 2010 il numero degli operatori del comparto bio è aumentato del 69 per cento, mentre gli ettari sono cresciuti del 79 per cento. Regioni come la Calabria, la Puglia e la Sicilia sono tra le prime a segnare questi incrementi. I nostri produttori di biologico sono avanti. Proprio per questo motivo, è essenziale l'approvazione di leggi come quella al nostro esame, perché sono segnali di vicinanza costante verso un comparto resiliente che porta in alto nel mondo il *made in Italy*.

Signor Presidente, onorevoli senatori, arriva oggi all'esame dell'Assemblea in modo inaspettato il disegno di legge che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Pur riconoscendo la necessità di dotare il Paese di un provvedimento tanto importante e atteso da anni, mi lascia molto perplessa la modalità con la quale oggi sia stato inserito all'ordine del giorno. Ormai sembra che si strozzi

il Governo per avere invece poi accolto la richiesta. Non credo sia giusto, anzi credo che sia molto grave. Per quanto mi riguarda devo sottolineare che quello che arriva in Aula oggi è un testo peggiorato e di certo non migliorato rispetto alla precedente versione. Il testo è stato modificato dalla Camera dei deputati, ma mentre si elimina dall'articolo 1 del testo in questione ogni riferimento al metodo biodinamico (riferimento per il quale si è sollevata tutta la società scientifica ed in modo particolare il Gruppo 2003,

Chiedo scusa, amici della Lega, sono sempre molto attenta quando voi parlate, invece mi pare che voi facciate sempre il contrario quando parlano gli altri. Si lascia invece all'articolo 5,

il metodo biodinamico dal tanto atteso provvedimento che avrebbe dovuto disciplinare il metodo biologico, ma si lasciano i rappresentanti al Tavolo tecnico, concedendo a questo metodo una corsia preferenziale e, cosa ancora più grave che potrebbe creare non pochi problemi, all'articolo 8, vale a dire in un momento delicatissimo di tutto il percorso quale è quello dell'adozione del Piano nazionale per le sementi biologiche, queste ultime non solo devono essere idonee al metodo biologico, ma anche evidentemente a quello biodinamico. Nel testo di legge, quindi, si verifica una contraddizione in termini, che pregiudica in due momenti fondamentali questo provvedimento: il valore e la e la trasparenza. Le discussioni in Commissione sono state lunghe ed accorate, e ringrazio per questo il Presidente e la Commissione tutta. Cito tra tutte la collega Silvana Abate, assente per motivi di salute, la quale ha sollevato con determinazione e argomentazioni giuridiche la gravosa questione, unitamente a me e alla senatrice Fattori. Ci uniamo sottoscrivendo l'ordine del giorno, preparato dall'autorevole senatrice Cattaneo, che già ebbe a presentare in prima lettura emendamenti abrogativi di ogni riferimento al metodo biodinamico agli articoli 1, 5 e 8 contenuti nel provvedimento in questione. Spero che l'ordine del giorno sia votato. Sarebbe un modo per dare voce anche a chi la pensa in modo diverso e che riesce a cogliere tra le righe i pericoli che si annidano in un provvedimento fondamentale e ritengo utilissimo per il futuro della comunità - parlo del biologico - che io personalmente

senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, siamo oggi chiamati ad approvare il disegno di legge inerente allo sviluppo e alla competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura Il settore dell'agricoltura biologica è in continua crescita e l'Italia rappresenta il terzo Paese europeo con oltre 2 milioni di ettari coltivati da 80.000 aziende. È una coltivazione che cresce di anno in anno e rappresenta il 16 per cento della superficie agricola utilizzata nel nostro Paese. I prodotti biologici sono molto richiesti ed è un mercato in continua crescita, incrementato dai consumi che aumentano ogni anno. In Italia il mercato di prodotti biologici ha un fatturato di 3,6 miliardi annui e il calo di importazioni da Paesi terzi ci permette di dare un maggior valore ai prodotti italiani,

Infatti, il 20 per cento dei giovani imprenditori agricoli si avvicina alla coltivazione biologica, che è considerata come concreta possibilità di ampliare le loro attività economiche, in particolare nei territori di collina e pedemontani, laddove l'agricoltura intensiva non è molto sostenibile, come avviene, invece, nei terreni pianeggianti. Ciò consente di valorizzare la tipicità dei prodotti locali e regionali, come è avvenuto nel Trentino Alto Adige dove, accanto alle numerose colture agricole, si sono promossi i distretti biologici, intesi come sistemi produttivi locali integrati a vocazione agricola, caratterizzati da una presenza significativa della produzione biologica. Si è provveduto, inoltre, alla tutela delle metodologie di allevamento e trasformazione tipica del luogo. La norma oggi in discussione può dare, quindi, un valore aggiunto alla nostra agricoltura, sostenendo i nostri prodotti a elevata qualità, che rappresentano la risposta moderna alle tradizioni locali che provengono dalle radici della nostra cultura e dall'identità dei nostri territori, ed è una legge che i nostri agricoltori ci chiedono da anni. La previsione, poi, del tavolo di filiera (qui all'articolo 16) per i prodotti biologici aiuterà nella promozione e nell'organizzazione di un mercato efficiente dei prodotti stessi e garantirà la stipulazione dei cosiddetti contratti di filiera. L'agricoltura biologica è considerata una tecnica di produzione privilegiata per il raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti. Tutto ciò avviene in un contesto ben preciso, in cui l'Unione europea, con il *green new deal*, la Farm to fork della biodiversità ha tracciato un orizzonte e un impegno preciso per la riduzione delle emissioni di gas serra, la salvaguardia della biodiversità e la creazione di un sistema di produzione del cibo meno impattante per l'ambiente. L'Unione europea conta inoltre di investire annualmente oltre 40 milioni di euro per promuovere il metodo dell'agricoltura biologica, intravedendo in questa tipologia di coltura uno strumento per accentuare e tutelare la salvaguardia della biodiversità, per un'agricoltura più sostenibile. Il piano d'azione prevede di sostenere i consumi, di aumentare di aumentare le produzioni biologiche in tutta Europa e di introdurre un nuovo regolamento per semplificare le procedure, rivisitare i controlli e rafforzarli per i prodotti biologici che arrivano da Paesi terzi. Quanto sopra si inserisce in un quadro più generale di politiche agricole e ambientali europee, finalizzato alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci e del 50 per cento della perdita di nutrienti del suolo, migliorandone la qualità. La proposta di legge oggi in argomento sottolinea come la produzione biologica sia un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di tutela della produzione alimentare; un metodo basato sull'interazione fra le migliori prassi in materia di ambiente, finalizzato alla salvaguardia delle risorse naturali e allo sviluppo ecosostenibile. Si tratta di metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari, applicati nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia

all'Assemblea due chiarimenti che ritengo necessari, visto che sul tema del biodinamico è stato detto di tutto e di più. È stato detto anche che regalavamo soldi all'esoterismo e cose del genere, quando nella norma non è previsto in alcun caso neanche un euro di erogazione a ciò che non è biologico. Ora bisogna intendersi: il biodinamico, così come è fatto in Italia, in tutti e tre i disciplinari che ne autorizzano la certificazione, prevede come obbligo

di nuovo riportata in due interventi in quest'Aula. Noi non stiamo parlando di una società economica - Demeter - che gestisce la materia. Questa è una fotografia di vent'anni fa. Oggi in Italia sono tre le società che fanno certificazione: oltre a Demeter, vi sono Agribiodinamica e Verdèa biodinamica, che egualmente certificano biodinamico,

solo informare l'Assemblea che i cosiddetti preparati biodinamici, di cui tanto abbiamo discusso e che sono l'oggetto del contendere sulle questioni esoteriche,

che sono stati recepiti nel nostro Paese da decreti ministeriali di recepimento dei regolamenti europei dal 1991 a seguire, quindi sono prodotti ufficialmente autorizzati all'utilizzo in agricoltura e in agricoltura biologica. Dico questo solo per chiarezza, altrimenti si ingenera la sensazione che stiamo parlando di chissà cosa: sono prodotti autorizzati dal 1991 nel nostro Paese. *(Applausi)*.

rispondere alle esigenze sia dei consumatori, sia dei produttori. Non a caso, proprio dal mondo agricolo, attraverso le rispettive associazioni di categoria, arriva l'appello ad approvare rapidamente il testo in esame. Si tratta infatti di un disegno di legge che risponde alle richieste del comparto agricolo e biologico, perché si pone l'obiettivo di difendere produttori e consumatori e di garantire la trasparenza degli acquisti, con misure concrete. Tra i diversi aspetti particolarmente qualificanti, si prevede ad esempio l'introduzione di un marchio *ad hoc*, che identifica come articoli al 100 per cento *made in Italy* soltanto i prodotti biologici ottenuti con materia prima nazionale. Inoltre, si potenziano i controlli e si favorisce l'uso di piattaforme digitali, per garantire una piena tracciabilità dei prodotti. Sono dunque tutte misure che mirano a difendere il comparto. Siamo contenti che con il voto di oggi si trovi un punto di mediazione, capace di superare la retorica secondo cui ci sarebbe contrapposizione tra agricoltura tradizionale, da un lato, e agricoltura biologica, dall'altro: il provvedimento in esame attesta che non è così; le coltivazioni biologiche si stanno rivelando un vero volano per il nostro *made in Italy*, al punto da rendere l'Italia il secondo Paese al mondo per volume di *export* di prodotti biologici, dopo gli Stati Uniti. un dato incredibile, se si confrontano le dimensioni dell'Italia con quelle degli USA. Tra l'altro, questa tipologia di coltivazioni ha il merito di favorire le Regioni economicamente più deboli, in particolare quelle del Sud, Sicilia, Calabria e Campania, che sono le prime per quantitativi di biologico prodotto, perché lì ci sono tra l'altro caratteristiche climatiche ottimali, che consentono un minore uso di fitofarmaci. Il biologico infatti non si può produrre ad ogni latitudine e il nostro Paese ha le condizioni climatiche e paesaggistiche più favorevoli, in un territorio che per il 70 per cento è collinare e montuoso. il biologico fa bene alle persone che ne fanno uso, fa bene ai territori nei quali si produce e fa bene ai produttori agricoli che lo coltivano. gli acquisti di prodotti bio *made in Italy*, ad esempio, hanno sfiorato il *record* di 7,5 miliardi di euro di valore, con 2 milioni di ettari di terreno coltivati. dimensioni che parlano da sole e che contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Farm to fork nel *green new deal* dell'Unione europea, che punta ad avere almeno un quarto della produzione agricola dedicata al bio anche nel nostro Paese. Ecco che per rispondere alle richieste che l'Europa ci pone sul *green deal* occorre agevolare la transizione al biologico da parte delle nostre aziende e per farlo servono norme *ad hoc*. Servono leggi come questa, questa, che ha il grosso merito di colmare quel vuoto normativo che fino ad oggi non ha consentito al settore di esprimersi in tutte le sue potenzialità. Gli indirizzi europei sono chiari e strumentalizzazioni varie su questo tema non trovano fondamento nella realtà di migliaia di imprese, imprese, che stanno consentendo a molti territori a rischio di abbandono non solo di continuare a vivere, ma anche di trovare nuove opportunità di sviluppo, in chiave moderna, sostenibile ed innovativa, con 80.000 imprese e un incremento dell'occupazione pari a ben il 71 per cento negli ultimi dieci anni, tanto che l'Italia è *leader* in Europa nel biologico. Si tratta dunque di un settore tutt'altro che minoritario, ma strategico, che rappresenta tra l'altro una quota rilevante del nostro *made in Italy*, sia in termini di mercato interno, sia a livello internazionale in termini di *export.* di *export.* È un settore che va sostenuto, soprattutto in un momento difficile come quello attuale. C'è da temere, infatti, che per l'agroalimentare italiano i prossimi mesi saranno ancora più duri di quelli passati per tanti motivi, a partire dall'aumento del costo del gasolio agricolo, passando per la mancanza di imballaggi, fino all'incremento spropositato del costo dei concimi e dei fertilizzanti: problemi veri, pesanti, che cadono sui nostri agricoltori, che adesso si dovranno confrontare pure con le nefaste conseguenze del conflitto in corso, anche alla luce delle diverse sanzioni adottate in questi giorni contro la Russia. Allora, signor Presidente, in un Paese come il nostro, nel quale negli ultimi anni è fortemente diminuita la superficie agricola coltivabile, dobbiamo dire con forza che servono più agricoltura e più modelli di agricoltura, compresa quella biologica, adatta a diverse condizioni climatiche e territoriali. Siamo convinti che il comparto agricolo sia un pilastro dell'economia del Paese e che vada sostenuto convintamente, con politiche di filiera che lo rafforzino. In particolare, proprio l'agricoltura biologica è un

Oggi più che in passato la scienza è di fondamentale importanza per affrontare la sfida della transizione ecologica, da un lato, ma anche per la modernizzazione dei processi produttivi, dall'altro, anche in ambito agricolo e può aiutare a coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale in un circuito virtuoso che punti a preservare il nostro modello produttivo agroalimentare, che è riuscito a fare della biodiversità e del rapporto con il territorio un vantaggio competitivo nel mondo. In questo modo togliamo anche ogni alibi a chi si oppone all'agricoltura biologica, accusandola di essere il primo passo verso la produzione di alimenti sintetici. Al contrario e lo ribadiamo ancora una volta - l'agricoltura biologica tutela il nostro modello di produzione agricola, non lo altera, lo protegge. Questo disegno di legge va nella direzione di rafforzare dunque un settore produttivo che fa del bene a tutto il nostro indotto agricolo e riconosce il lavoro, l'impegno, la dignità e anche la resilienza di un comparto, quello biologico, importante per lo sviluppo sostenibile del Paese. Per concludere, signor Presidente, vorrei ribadire anche quanto siamo orgogliosi di tutti i nostri produttori agricoli, persone che fanno un lavoro anche fisicamente molto duro, esposto più di altri a variabili climatiche ed economiche. Desidero esprimere la nostra gratitudine per i tanti prodotti di grande eccellenza che riescono a offrire, prodotti che così frequentemente ci rendono famosi in tutto il mondo. mondo. Voglio ringraziarli anche per aver saputo garantire con grande fatica e con grande sacrificio l'approvvigionamento delle nostre tavole nei momenti più duri del primo *lockdown* e della pandemia. Insomma, signor Presidente, penso che il voto di oggi sia una bella pagina per il nostro Paese, perché approvare questo provvedimento vuol dire fare l'interesse di tutta la nostra società e di un'economia reale in vera crescita. crescita. Nel ringraziare dunque il relatore Taricco, il Presidente della Commissione agricoltura e i colleghi tutti, nonché la Presidenza del Senato per aver voluto calendarizzare il provvedimento celermente, dichiaro con piacere il voto favorevole del mio Gruppo. [LA

l'importanza dell'agricoltura, ma - mi rivolgo al Governo e ai colleghi di maggioranza - al di là delle parole di tutti i complimenti che facciamo ai nostri agricoltori e ai nostri allevatori, sarebbe opportuno essere anche più concreti, perché fondamentalmente la concretezza si misura anche con quante risorse il Governo mette a disposizione dell'agricoltura. Purtroppo nei vari provvedimenti che abbiamo visto, dalla legge di bilancio al PNRR, queste risorse non sono adeguate, né all'altezza di questo questo comparto che è definito primario, ma che è fondamentale anche per la nostra economia. Il disegno di legge che oggi finalmente ci accingiamo ad approvare in quarta lettura in maniera definitiva è sicuramente un passo importante, una legge quadro, quadro, di fatto, che mette ordine al comparto della produzione biologica nella nostra Nazione, perché, com'è già stato sottolineato e come abbiamo già detto tante volte nelle varie dichiarazioni di voto e nei vari interventi che abbiamo fatto anche nelle letture precedenti, è un comparto importante

concentrare l'attività dell'agricoltura interamente sul settore del biologico, perché come sappiamo l'agricoltura biologica ha

a tutti i cittadini di potersi alimentare in maniera corretta, perché non possiamo comunque pensare di avere poi cittadini di serie A e di serie B, che, in base alle loro possibilità economiche, possono alimentarsi meglio o peggio rispetto ad altri. Questo è un ragionamento di carattere sociale molto importante, che mi sta particolarmente a cuore. quindi che questo disegno di legge abbia regolarizzato tutto il comparto, ma stiamo attenti a questi aspetti. Oggi, purtroppo, la situazione che è scoppiata in Ucraina, la guerra che qualcuno di voi ha già citato, ci porta ad una riflessione per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare del nostro Paese, perché non c'è soltanto un problema legato all'energia, ma ne abbiamo anche uno che dovremo affrontare e su cui dovremo confrontarci per quanto riguarda l'autosufficienza alimentare. dall'Ucraina e dalla Russia arriva circa il 25 per cento del grano duro che importiamo: capite che questo, insieme anche alle politiche agrarie del Canada, degli Stati Uniti dell'Australia, incide pesantemente anche sui costi, ma fondamentalmente ci deve portare a riflettere su quanto stiamo facendo nel nostro Paese per raggiungere l'autosufficienza alimentare, perlomeno in certi settori. Noi purtroppo non l'abbiamo in nessun settore, ma non esiste non esiste oggi un piano strategico nazionale per la sicurezza alimentare. Su questo dovremmo confrontarci e dobbiamo investire risorse e avere sicuramente una visione, tutti uniti per i prossimi anni. Detto questo, vorrei però anche mettere in chiaro alcune cose che sono successe nell'*iter* di questo provvedimento. Peraltro, sono contento che la che la senatrice Cattaneo abbia accettato le riformulazioni proposte dal Governo, perché anche da qui nascono un atto unanime e un impegno affinché si possano correggere le sfumature che ancora rimangono nel disegno di legge. Come Fratelli d'Italia,

però sempre combattuto l'equiparazione che c'è all'interno della legge tra biodinamico e biologico, tant'è che in seconda lettura avevamo proposto in Commissione agricoltura degli emendamenti per l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1, che sono stati bocciati.

In quell'occasione, la senatrice Cattaneo presentò emendamenti su cui noi, coerentemente con la linea che avevamo avuto in Commissione, abbiamo espresso voto favorevole. è andato alla Camera ed è stata fatta una modifica all'articolo 1, ma purtroppo - com'è già stato sottolineato - all'articolo 5, che riguarda il tavolo tecnico del Ministero per il biologico, e all'articolo 8, che riguarda il piano nazionale,

il biodinamico e poi farlo rientrare della finestra, facendo partecipare un rappresentante di questa categoria al tavolo tecnico, e riconoscerlo anche all'interno del piano nazionale per le risorse che devono essere distribuite. Come dicevo, sono soddisfatto del fatto che la senatrice Cattaneo abbia presentato quest'ordine del giorno e abbia accettato le riformulazioni, perché è chiaro che c'è un impegno preciso del Governo a far sì

opera nel nostro Paese ed era in attesa, dopo tutta una serie di tentativi in tutte le legislature che ci hanno preceduto, che fosse varata una legge sull'agricoltura biologica. Con il voto odierno mettiamo in campo questo strumento importante. risolutivo dei problemi dell'agricoltura, che sono tuttora tanti e ne abbiamo tanti all'orizzonte, ma sicuramente per il comparto è una risposta assolutamente importante. È un giorno di festa

è stato detto che c'era come riferimento unico un'azienda privata e non è vero, perché sono tre i soggetti che fanno certificazione; è parlato dei preparati biodinamici, che, come dicevo prima, dal 1991 sono legalmente autorizzati dall'Unione europea e dai decreti ministeriali italiani di attuazione. Si è detto che quel termine, biodinamico, portava l'equiparazione. Ricordo solo i documenti disponibili a tutti coloro che, oltre a parlare, vogliono provare anche a leggere le cose che vi stanno scritte: quel termine è arrivato dalla Camera, perché il termine biodinamico lo abbiamo ricevuto da lì; è agli atti, alla Camera e al Senato,

Oggi, con la norma vigente, quel riferimento al biodinamico è controllabile, in quanto biologico, soltanto in virtù dei propri disciplinari, mentre, mettendolo in legge, lo era in virtù di legge. Devo dire che, da questo punto di vista, il testo che rimane approvato non toglie nulla all'efficacia dei controlli, perché di fatto, al comma 3 dell'articolo 1 reca: «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica». Dato che la produzione biodinamica utilizza preparati riconosciuti dall'Europa e dai decreti ministeriali e ha nei propri disciplinari produttivi l'obbligo di certificazione biologica, a tutti gli effetti rientra in questo articolo. Credo che queste puntualizzazioni fossero necessarie. Mi rimane una sorta di retropensiero: che si sia voluto attaccare sul cornoletame e su altre questioni per non parlare del biodinamico e di ciò che è realmente. Il biodinamico

Il metodo biodinamico centra la produzione sulle rotazioni, sui sovesci e sull'attenzione all'*humus* nel terreno, obbliga rotazioni con terreno lasciato a riposo per sostenere

Il fatto che oggi invece siamo qui per approvare la legge sul biologico è un dato molto importante, perché il biologico è per il nostro Paese una ricchezza straordinaria. Cito solo due dati: in Italia ci sono 2 milioni di ettari oggi coltivati a biologico, con oltre 80.000 operatori del settore in crescita, con il 16 per cento dell'agricoltura, 4,6 miliardi di consumo interno, in crescita rispetto all'anno scorso del 5 per cento, e con una spesa per le famiglie che, a parità di produzione, è cresciuta del 133 per cento nell'ultimo anno. Gli ultimi sondaggi dicono che nove famiglie su dieci hanno fiducia nel biologico e che una su due, quando può ed il prezzo è accessibile, compra biologico.

devono essere di grande soddisfazione per tutti noi. Abbiamo reso un servizio importante all'agricoltura e al nostro Paese. Voglio essere molto chiaro. Credo che abbiamo all'orizzonte - e l'impegno della Commissione agricoltura a questo è sempre stato dedicato di affrontare e risolvere tutti i problemi di tutte le forme di agricoltura, valorizzando tutte le potenzialità che ci sono. Al riguardo non c'è alcuna discussione. Credo però che, proprio perché abbiamo tale obiettivo, questo segmento, destinato a diventare un quarto dell'agricoltura del nostro Paese e dell'Europa, debba essere valorizzato. Ritengo che con il passo di oggi diamo un sostegno importante nella giusta direzione.

Il tema dell'agricoltura biologica è oggi, ancora più di ieri, assolutamente centrale e fondamentale per il nostro Paese. Dobbiamo chiarirci una volta per tutte. Si tratta di un tema centrale per il processo di

25 per cento. L'Italia da questo punto di vista è il Paese che ha investito di più,

che la nostra agricoltura non è unica, ma che ci sono tante agricolture legate al territorio. Questo è il nostro vantaggio, su cui in questi anni abbiamo lavorato per far sì

non pensate che la lotta ai cambiamenti climatici - di cui l'agricoltura è uno degli elementi centrali - si faccia solo e unicamente con la transizione energetica. Si fa anche, per esempio, non impoverendo più i nostri suoli,

di pensare che l'agricoltura biologica sia quella dei figli dei fiori o dell'improvvisazione, perché è basata su metodi

- le nostre tecniche di coltivazione. Colleghi, non sono un'integralista, però penso che proprio dall'agricoltura biologica arrivino tanti insegnamenti e abbiamo bisogno di più scienza

a mettere in campo gli strumenti che servono ai nostri produttori, sapendo che abbiamo avuto e abbiamo un vantaggio competitivo. Abbiamo avuto indicatori

per cui il consumatore, il cittadino, ha ben compreso quanto sia importante per l'ambiente, per gli ecosistemi e per la propria salute cominciare o continuare a consumare bio.

perché sono gli interessi della nostra agricoltura, del nostro Paese, degli ecosistemi e della salute dei cittadini. Signor Presidente, cari colleghi, con il voto di oggi sul disegno di legge sul biologico abbiamo finalmente l'occasione di portare l'agricoltura italiana nel XXI secolo.

che equiparava, sin da allora, il biologico al biodinamico. Oggi la senatrice Bonino ha cambiato idea, ma gli eventi tragici cui stiamo assistendo ci dimostrano che la transizione verso uno sviluppo più sostenibile è una necessità che non possiamo più rinviare. In questo contesto, anche una misura destinata al settore agricolo può dare un contributo prezioso al cambiamento di cui avvertiamo urgente bisogno.

Pur in assenza di uno strumento normativo nazionale, l'Italia, attraverso gli strumenti di mercato, è riuscita a raggiungere obiettivi considerevoli: è la quarta per produzione in Europa, per superfici coltivate e per numero di produttori. Le produzioni bio rappresentano quindi una punta di eccellenza del sistema agroalimentare italiano, nel quale Forza Italia crede fermamente, sostenendo gli imprenditori impegnati in questo comparto. *(Applausi)*. È un *trend* di mercato in continua ascesa, con circa 2 milioni di ettari e oltre 80.000 aziende. Nel 2020 il fatturato di questo mercato, come hanno detto anche altri colleghi, ha raggiunto quote di 7 miliardi di euro, con un incremento del 142 per cento dal 2010. Il consumo interno è inarrestabile. Sono ottimi risultati, ma siamo convinti che si possa fare molto di più, anche grazie al presente disegno di legge. Il nostro Paese è infatti naturalmente vocato in Europa a questa concezione dell'agricoltura. In particolare, il Mezzogiorno ha una vocazione che rende la Sicilia, la Calabria e la Puglia le aree elette per la produzione di prodotti biologici e biodinamici.

le rotazioni e il minor fabbisogno di *input* energetici e chimici mettono al riparo dagli *shock* inflattivi e dalla scarsità di mezzi tecnici necessari all'agricoltura intensiva. mattina alcuni agricoltori della Coldiretti intervistati lamentavano proprio la difficoltà di concimare i loro seminativi per l'impennata dei prezzi dei concimi e dei diserbanti. Bene: un'agricoltura biologica, con la concimazione

più confortevole, più utile e più favorevole a tutto il sistema Paese. *(Applausi)*. I distretti del bio, la possibilità di registrare il marchio biologico *Made in Italy*, la razionalizzazione dei controlli e altri meccanismi contenuti nella norma possono davvero agevolare l'ulteriore espansione di un settore che, come ho detto, incontra il favore dei consumatori, in Italia e all'estero. Ciò che bisogna garantire, però, è che il biologico non diventi appannaggio di pochi soggetti elitari, più forti, ma costituisca realmente un nuovo metodo di produzione e di impresa diffuso, che vada a beneficio dei produttori e di quelle comunità rurali che oggi vedono nell'abbandono della terra l'unica possibilità per evitare un grave accumulo di perdite. Come Italia abbiamo davvero l'occasione di farci capofila in Europa di questo rilancio del settore primario tra le altre cose, anche di garantire l'autonomia di approvvigionamento e di produzione, che in questi giorni abbiamo visto essere un tema fondamentale degli equilibri nazionali ed internazionali. L'Europa ha bisogno di un cambio di paradigma, che può partire dal settore primario e indicare quella strada al resto dell'economia, senza però discriminare nessuno. Abbiamo visto come l'aver escluso il riferimento esplicito al biodinamico dagli articoli 1 e 21 non dovrebbe cambiare granché, perché la biodinamica non è una *lobby,* ma una branca rigorosa del metodo biologico, come è stato detto anche di cui però rispetta tutte le norme. Non ci saranno, dunque, problemi ad ottenere le incentivazioni. I produttori possono stare tranquilli, potranno continuare a produrre anche coltivazioni biodinamiche in Italia,

Vorrei ricordare che l'agricoltura biodinamica, senatrice Cattaneo, è già contenuta nella legislazione europea: i regolamenti europei sul bio furono mutuati proprio dai disciplinari biodinamici

La biodinamica, dunque, cari colleghi, non è una novità di questo disegno di legge: quando c'è una caccia delle streghe, è dagli inquisitori che bisogna difendersi.

il biologico è un tema importantissimo per il nostro Paese, ma io vorrei ricordare i numeri della nostra agricoltura, che vale quasi 32 miliardi di euro;

di legge è importante e si inserisce in un contesto di grande difficoltà per l'agricoltura italiana. Direi che oggi è anche un momento di grande festa per inaugurazione della fiera agricola di Verona, un evento straordinario a livello internazionale, dove sicuramente ci saranno delle attrezzature, ci saranno dei momenti informativi e di comunicazione in merito soprattutto all'agricoltura biologica.

dia la possibilità di produrre cibi genuini. Nella difesa di questa agricoltura noi andiamo a cercare anche la difesa della salute del consumatore, che è fondamentale. Nell'ultimo decennio le vendite di prodotti biologici sono cresciute di oltre il 122 per cento, una cifra importante; il successo dei consumi sostiene l'aumento della produzione che c'è nel nostro Paese, come è stato detto prima dai colleghi. Siamo i primi produttori europei e siamo i secondi al mondo, ma con una capacità di controllo del prodotto che solo l'Italia ha a livello europeo e a livello mondiale. Questo lo dobbiamo riconoscere al nostro settore dell'agricoltura, ma soprattutto lo dobbiamo riconoscere ai nostri produttori, che faticano e vivono anche una pratica burocratica che, attraverso questo provvedimento, cercheremo di

di pieno fermento del settore si inserisce il disegno di legge in esame, che può quindi dare un contributo importante a tutto questo nostro mondo. Tra i punti maggiormente qualificanti - lo voglio ricordare - il provvedimento prevede l'introduzione

Nel biologico c'è infatti - lo dobbiamo dire anche rispetto all'*italian sounding* e a tutte le contraffazioni del prodotto italiano nel mondo nel mondo - un vero e proprio allarme per l'invasione di prodotti da Paesi extracomunitari, con un incremento della quantità di prodotto di oltre il 10 per cento annuo e con circa un terzo dei prodotti provenienti dall'Asia, c'è una difficoltà di controllo molto elevata, come abbiamo potuto verificare nelle audizioni svolte in Commissione agricoltura. Il marchio poi rappresenta uno strumento importante per rafforzare la presenza dei prodotti nazionali sui mercati esteri. È stato fatto molto

con molta attenzione all'innovazione, soprattutto nel mondo dei giovani. Il disegno di legge prevede infatti la possibilità di creazione di piattaforme digitali per garantire una piena informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti, con una delega al Governo - e qui ritorna in campo l'attività dei nostri Ministri e dei nostri Sottosegretari - per rivedere la normativa sui controlli e garantire l'autonomia degli enti di certificazione. Elementi importanti vengono introdotti nella legge anche per la definizione e il riconoscimento dei biodistretti, come anche si introducono nel nostro ordinamento delle forme di rappresentanza adeguatamente riconosciute e valorizzate (cosa che oggi mancava), innovative per il biologico, in quanto finora previste solo per altri specifici settori. auspicio è quello di contribuire a sostenere con questa legge un sistema più grande, quello dell'agroalimentare nazionale, per il quale possono aprirsi nuove prospettive di sviluppo, rendendolo appetibile alle giovani generazioni e facendo in modo che ci sia una redditività,

Dall'altra parte abbiamo il problema della peste suina africana, che non è stata assolutamente debellata; anzi, siamo in fase di discussione del relativo provvedimento. C'è inoltre la problematica

che nel frattempo si riesca a dare forza ed energia alle altre misure per aiutare il comparto agricolo e agroalimentare italiano, sempre nella visione di un consumatore attento soprattutto alla sua salute. *(Applausi)*.

due modifiche lo scorso 9 febbraio, che abbiamo poc'anzi accolto, con voto favorevole. Le due modifiche appena apportate riguardano l'articolo 1 e l'articolo 21 La modifica intervenuta all'articolo 1, comma 3, ha di fatto eliminato l'esplicita equiparazione dell'agricoltura con metodo biodinamico a quella biologica, lasciando una generale possibilità di equiparazione con il metodo biologico a quelle forme di agricoltura che ne seguono i protocolli disciplinari. Ringrazio il senatore Taricco per il grande lavoro fatto e per lo spirito di verità che ha messo nel suo intervento e nelle sue precisazioni puntuali, quali quelle sui regolamenti comunitari sul biologico, recepiti da decreti ministeriali, che già dal 1991 - quindi da trenta anni - consentono l'uso di preparati biodinamici nei metodi biologici. Abbiamo accolto l'ordine del giorno della senatrice Cattaneo, perché, pur espungendo ulteriormente il biodinamico da questa normativa, nei fatti il biodinamico resta nel biologico a pieno titolo. La seconda modifica è intervenuta sull'articolo 21, estendendo anche ai decreti legislativi di attuazione delle disposizioni previste dal disegno di legge la loro applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il testo nel suo complesso costituisce una legge di riferimento per l'agricoltura biologica, invocata da diverso tempo, la cui stesura ha richiesto molteplici accorgimenti, per rispondere alle tante istanze giunte dagli operatori del settore. tema importantissimo, in quanto occupa posti di rilievo in Europa e nel mondo, sia per superficie coltivata, sia per numero di imprese che operano nel settore. Tutto ciò avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il *green new deal* e con il Farm to fork, si pone l'obiettivo di arrivare, nei prossimi anni, cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica, investendo oltre 40 milioni di euro nella sua promozione, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. Lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione su tutto il territorio d'Europa. questo si inserisce quindi all'interno di un quadro generale di politiche agricole e ambientali, che punta alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci, del 50 per cento della perdita di nutrienti nei suoli e del 50 per cento dell'utilizzo di antimicrobici che oggi approveremo definisce il concetto di agricoltura biologica, in gran parte mutuandolo da regolamenti comunitari. Si definisce il ruolo che svolgeranno le Province e le Regioni, si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico e l'istituzione di un marchio dell'agricoltura biologica, per un messaggio chiaro, che generi valore ed economia, che parli di rispetto della natura e della salute, di semplicità, di ritorno alla genuinità e alle tradizioni, di attenzione in ogni fase della lavorazione. Si prevede un piano d'azione nazionale, sia per la produzione biologica che per i suoi prodotti, adottato a cadenza triennale, con l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico e sostenere la costituzione di forme associative, che aiutino le imprese agricole, anche favorendo nuovi insediamenti e migliorandone il sistema di certificazione e di controllo. È previsto anche un piano nazionale delle sementi biologiche, sostenendone la ricerca, come per tutte le pratiche innovative. È fondamentale, per l'agricoltura biologica, che non si tratti di un tema di singole aziende, ma sia esteso ai territori: da qui l'istituzione dei distretti biologici, al fine di snellire le certificazioni, considerandole a livello di territorio. Viene affrontato tutto il tema del riconoscimento e della disciplina delle filiere, caratterizzandole proprio su questo tipo di aziende. Riguardo alla questione importante dei controlli è data delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle normative. Abbiamo nelle nostre mani una vera e propria legge quadro, che crediamo possa mettere in condizione il settore di raggiungere obiettivi ambiziosi, per ridurre l'utilizzo di fitofarmaci, per aumentare la resistenza delle colture agricole e la fertilità del suolo e, quindi, per una maggiore resilienza al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Lavorare dunque la terra con il metodo biologico significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetti i cicli vitali naturali. Dopo anni di utilizzo di sostanze chimiche e di sintesi, ci troviamo con pochissima sostanza organica nei suoli e con una preoccupante presenza di residui di fitofarmaci nelle acque. quindi indispensabili norme rigorose di produzione, che contribuiscano al rispetto dell'ambiente, da cui deriva la qualità dei prodotti, nonché il benessere degli animali. Il consumatore vuole mangiare sano e in modo etico ed è un valore anche l'italianità del prodotto. Tutto il mondo invidia la nostra cucina e le materie prime che crescono nei nostri campi, maggiormente se contraddistinte da marchi di garanzia e di qualità a tutela a tutela del consumatore. Se c'è davvero una nuova consapevolezza sull'importanza del suolo agricolo e del suolo naturale, oltre che di un ambiente nel suo complesso non inquinato, è ora di dimostrarlo con politiche indirizzate a questi scopi. L'agricoltura biologica è una delle possibilità concrete che abbiamo. Per questo, per le ragioni che ho illustrato, dichiaro convintamente il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

può un'azienda con un fatturato di oltre 8 miliardi di dollari permettersi il taglio al personale? Purtroppo in Italia pare di sì. È quanto sta succedendo a Catania, in Sicilia, e l'azienda interessata è una multinazionale conosciuta in tutto il mondo

marzo i lavoratori e i sindacati locali faranno una manifestazione chiedendo chiarezza, perché non hanno certezza delle prospettive.

dei lavoratori e lavora nell'ambito delle produzioni asettiche. Il particolare strano è che il 7 febbraio è stata consegnata alle rappresentanze sindacali una comunicazione per una procedura di riduzione del personale, ma il 3 febbraio, dopo un lungo silenzio durante il quale era avvenuta la dismissione di un compartimento produttivo penicillinico, l'azienda ha comunicato che avrebbe intrapreso una procedura di riduzione del personale, pur avendo stanziato 26 milioni di euro per degli investimenti nel sito, una quota che però non sarebbe sufficiente agli adeguamenti richiesti dall'Annex 1, linee guida emanate dagli enti regolatori per la produzione dei farmaci. con tale intervento si richiede un'immediata soluzione, un tavolo tecnico con il Ministero, di concerto con la Regione Siciliana, e possibilmente anche un'immediata risposta

Presidente, se c'è violenza, non ci può essere amore. L'amore presuppone il rispetto per l'identità dell'altra persona, per la sua libertà, comprende la gioia per la realizzazione dell'altro. Nessuno può essere oggetto di possesso da parte di un'altra persona, il possesso non è amore. Annullarsi per l'altro non è amore. Quando non si accetta l'autonomia dell'altra persona, il rapporto diventa asimmetrico e doloroso. Ecco che allora per alcuni soggetti il rifiuto, la separazione dal *partner* scatena comportamenti liberticidi, frutto di una cultura arcaica di uomini che non sopportano che la donna sia realizzata ed emancipata, persino che sia felice. nella nostra società tutto ciò avviene nonostante i diritti acquisiti e le pari opportunità che la Carta costituzionale garantisce. Ecco che allora non è raro che l'abbandono di un uomo da parte di una donna scateni la violenza, la violenza, che a volte sfocia in femminicidio, che altro non è che l'omicidio di una donna per il solo fatto di essere donna, al fine di sopprimere i suoi diritti, perfino la sua felicità. A dicembre 2021 sono state uccise in ambito di relazioni familiari o affettive 98 donne, di cui 66 hanno trovato la morte per la mano del *partner* o dell'ex *partner.* Dunque l'assassino in genere ha le chiavi di casa, ma purtroppo non sempre i casi di violenza domestica si riescono a intercettare per tempo, nonostante in genere il femminicidio sia solo la conclusione di un'*escalation* che inizia con reati minori quali i maltrattamenti in famiglia, *stalking*, minacce, lesioni. È quello che è accaduto la settimana scorsa in Sardegna, a Porto Torres, dove un muratore di Ploaghe ha ucciso a colpi di accetta il suocero, un ex poliziotto, e ferito gravemente la moglie e la suocera sotto gli occhi di due gemellini. caso, si è trattato di un duplice tentato omicidio. Ricordiamo, Presidente, che la recente riforma Cartabia è intervenuta sul punto colmando una profonda lacuna del codice rosso. L'articolo 2, infatti, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. In particolare, la portata applicativa di alcune disposizioni del codice di procedura penale a tutela delle vittime, che è attualmente limitata ad alcune fattispecie delittuose (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori, lesioni personali), è stata estesa alle vittime dei...

vorrei portare l'attenzione su un tema che interessa direttamente la Regione Campania e precisamente la località di Persano, nel Comune di Serre, in provincia di Salerno, e che riflette i suoi effetti sulla credibilità del nostro Paese nelle relazioni internazionali, ma soprattutto sull'impatto ambientale di scelte scellerate. Si tratta della vicenda relativa a 7.900 tonnellate di rifiuti che la Tunisia ha rispedito al mittente dopo aver asserito che dall'Italia erano partiti oltre duecento *container* contenenti rifiuti indifferenziati misti a rifiuti ospedalieri. In conseguenza del presunto comportamento illecito delle ditte italiane che hanno trattato e spedito i rifiuti dall'Italia alla Tunisia, le autorità tunisine hanno aperto delle indagini a seguito delle quali la Regione Campania ha stipulato un'intesa per il rientro dei rifiuti in Italia. Dal 22 febbraio scorso questi rifiuti di dubbia provenienza stazionano nel porto di Salerno e il rischio di un disastro ambientale in Campania è ancora una volta dietro l'angolo. Le associazioni ambientaliste hanno provato in ogni modo possibile a fermare il rimpatrio di questi rifiuti di dubbia provenienza, ma purtroppo il peggio non è stato in alcun modo scongiurato, nonostante i sigilli dei *container* apparissero manomessi e non vi fosse alcuna certezza riguardo al loro contenuto. A completare il quadro già di per sé drammatico è la scelta della destinazione finale di questi *container*, che verranno trasferiti in località Persano, nel Comune di Serre, in provincia di Salerno, in vista del loro avvio a smaltimento e recupero presso ulteriori destinazioni. Il sito in questione è ubicato all'interno di un'area naturalistica di alto pregio ambientale, l'oasi WWF di Persano in Salerno, cosiddetta zona umida di importanza nazionale caratterizzata dalla presenza di ambienti naturali incontaminati. Ancora una volta, a pagare le spese della negligenza saranno territori di alto valore geologico. La piana del Sele e la Regione Campania non sono non sono purtroppo nuove a tali disastri. Per questo oggi mi trovo costretta ad appellarmi a tutte le istituzioni coinvolte, affinché si tuteli quando più possibile questo territorio da danni ambientali inestimabili

Alla ASL Roma 3 si riscontra una grave carenza di neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, assistenti sociali e logopedisti, con ripercussioni gravissime non solo sulle famiglie ma anche sui docenti. Queste figure

salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva. A seguito, quindi, delle sollecitazioni del comitato, che ringrazio, promotore del servizio di neuropsichiatria infantile della ASL Roma 3 e dei Gruppi

a livello nazionale, è noto che, con il decreto sostegni-*bis* abbiamo stanziato circa 20 milioni per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e di adolescenza,

La dottoressa Antonia Giammaria, pubblico ministero di Roma, già vice capo gabinetto dell'ex ministro Calenda, che avrebbe avuto il dovere di comportarsi con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nello svolgimento del suo ruolo, al contrario, come si può leggere anche nel ricorso al TAR del Lazio del Codacons e contestuale richiesta di equa riparazione alla procura della Corte d'Appello, sembra abbia svolto il suo ruolo in maniera arbitraria. Per aver presentato un'interrogazione, il 17 luglio 2018, sulla nomina del dottor Capecchi a direttore Agcom, ricevevo un avviso di garanzia, per reato di cui all'articolo 595 del codice penale, firmato l'11 settembre 2018 dalla dottoressa Giammaria. Convocato il 25 settembre 2018 da un solerte ufficiale della Guardia di finanza, che lavorava alla stessa Agcom di cui il dottor Capecchi era direttore generale, alla presenza del mio avvocato, Francesco Strigari, ribadivo che l'atto di sindacato ispettivo rientrava nelle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione. Il procedimento penale doveva, quindi, essere archiviato in tempi ragionevoli. Ciononostante, il pubblico ministero Giammaria chiedeva proroga delle indagini. Il 20 luglio 2021, a quasi due anni dalla scadenza del termine della proroga, l'avvocato Strigari presentava istanza di sollecito, chiedendo alla Giammaria di promuovere al gip la richiesta di archiviazione per insussistenza di reato e per l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Diritto di critica e dubbi si evincevano dal *curriculum*, scritto di pugno dal Capecchi stesso e pubblicato in rete. Interesse pubblico dei cittadini italiani e continenza: le forme da me utilizzate in quella interrogazione erano pacate e limpide, i toni mai offensivi né scurrili. Il 30 luglio 2021 reiterava seconda istanza di sollecito; il 26 ottobre la terza istanza. Solo il 17 ottobre la pubblico ministero Giammaria chiede finalmente che il gip voglia disporre l'archiviazione del procedimento, dopo aver osservato che, dall'esame degli atti, non sono emersi elementi che permettano di configurare le ipotesi di reato ascritte e che non sono stati indicati altri elementi di sufficiente spunto investigativo. Ne consegue che, per le esposte considerazioni, si deve avere Il giorno dopo, il 18 ottobre, dunque a 3 anni e un mese dall'avviso di garanzia, il giudice per le indagini preliminari, Patrone, letta la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero, ritenuto che la motivazione della richiesta è pienamente condivisibile, alla luce degli atti presentati dispone l'archiviazione.

benché senatore, appeso per 37 mesi sotto la spada di Damocle di un reato inesistente, merita di essere duramente sanzionato da un CSM, il cui grave scandalo disonora l'intero ordinamento giudiziario, minando irrimediabilmente la residua fiducia nella giustizia. Io mi auguro che d'ora in avanti i pubblici ministeri, quando si invoca l'articolo 68 della Costituzione, non tengano per tre anni i senatori e i deputati appesi